L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della

Gentili senatrici, gentili senatori, domani, venerdì 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza che tocca i cuori e le coscienze di tutti.

che, assieme alla presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello, al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, all'ambasciatore d'Israele in Italia Alon e a tanti altri esponenti della comunità - mi scuso se non posso citarli tutti - ci onorano qui oggi con la loro presenza: una presenza tanto importante quanto significativa che salutiamo con un caldo e affettuoso applauso.

così rilevante, che io stesso, da Presidente del Senato, ho proposto ai Gruppi parlamentari registrando una totale adesione, possa contribuire ad arricchire le iniziative e le opportunità che tutti insieme dobbiamo mettere in campo affinché il ricordo dell'immane tragedia della Shoah possa essere sempre più memoria condivisa di una comunità nazionale che ripudia con forza ogni forma di odio, di discriminazione, di razzismo, di antisemitismo e di antisionismo

nella Sala della Costituzione a Palazzo Giustiniani, dove ha portato la sua testimonianza agli studenti del liceo «Morgagni» di Roma. In quell'occasione ho voluto non esserci proprio per non dare neanche il minimo accenno di politicizzazione di un tema che deve appartenere a tutti. Ringrazio Modiano per essere venuto.

Il Senato della Repubblica è stato e sarà sempre in prima linea per diffondere il significato di questo giorno. Quest'anno lo abbiamo voluto celebrare in forma ancora più più solenne. Tutti noi abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere, soprattutto alle generazioni più giovani - lo sottolineo - il dramma e le atrocità che subirono gli ebrei a partire dall'infamia delle delle leggi razziali italiane. È compito di tutti, a cominciare dalle più alte istituzioni, tramandare il ricordo affinché in futuro non si ripetano mai più simili tragedie; il modo migliore è quello, appunto, della memoria: senza la memoria non c'è mai la certezza che non vi sia la ripetizione di gesti odiosi. È necessario guardare al presente e al futuro con la doverosa attenzione verso ogni forma di razzismo e di antisemitismo, che non può e non deve mai più trovare cittadinanza 2008 ero Ministro della difesa e fui il primo Ministro a recarmi, Pacifici (anche lui qui presente, lo saluto, lo ricorderà), a rendere omaggio ai caduti ebrei della Prima guerra mondiale, a italiani ebrei che erano morti difendendo

potrebbe sicuramente pensarci. A proposito, oggi il Senato, col suo concorde e unanime momento di riflessione e di memoria, vuole indicare a tutti la necessità di non fermarci alla solennità, proprio perché lo facciamo in maniera solenne. Vorremmo che il Giorno della Memoria entrasse nella quotidianità,

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, non importa quanto sia buio il presente, si può sempre illuminare il futuro. Così scriveva la piccola Anne Frank negli anni in cui, con la sua famiglia, era costretta a nascondersi in un sottotetto, per sfuggire alla follia generata dall'odio che poco più di settant'anni fa ha travolto l'Europa e il mondo intero, sconvolgendo una generazione intera, dalla quale è nostro onore e onere raccogliere il testimone della memoria. È commovente pensare come una ragazzina di appena quattordici anni, alla quale era stata rubata di colpo l'infanzia, la spensieratezza della giovinezza, non avesse perso, nonostante tutto, la capacità di sperare. È su quella speranza che negli ultimi decenni si è cercato di costruire una consapevolezza comune. L'Olocausto rappresenta una macchia indelebile nella storia dell'umanità che non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare, come ha appena ricordato il presidente La Russa. La libertà non va mai data per scontata, amici; abbiamo imparato perché avevamo anche dimenticato che potesse esserci la guerra alle nostre porte e invece, come abbiamo visto, purtroppo non possiamo fare a meno di prenderne appunto, è una macchia indelebile e non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Solo attraverso la memoria e il ricordo vivo, costante e sincero si potrà evitare che fatti tanto orribili possano verificarsi nuovamente, perché se è vero che la società di oggi è più consapevole, è anche vero che non sono infrequenti episodi di odio e discriminazione anche tra i più giovani, che devono essere stigmatizzati e non sottovalutati. Il senso della giornata che ci troviamo a celebrare nella sede della più alta istituzione parlamentare del nostro Paese ricordare e onorare. Va detto, però, che il ricordo non è e non deve essere fine a se stesso; anzi, al contrario il ricordo deve essere considerato uno strumento della più importante finalità che ha portato all'istituzione di questa giornata: la prevenzione. Se così non fosse, si finirebbe per trattare l'Olocausto come un semplice episodio della storia, destinato ad essere studiato, magari al più approfondito, oggetto di qualche sceneggiato televisivo il 27 gennaio, ma destinato a cadere nell'indifferenza emotiva, come ha sottolineato in questi giorni la senatrice Segre. Mi riferisco proprio a quella stessa indifferenza che ha dato origine a quei fatti riprovevoli che accadevano anche nel nostro Paese, a fianco alle nostre case. Penso a Bolzano, la mia città, che proprio nell'anno appena concluso è stata la città della memoria, dove venne costruito un campo di concentramento, che i più non conoscono, famoso forse solo perché vi è stato prigioniero per quindici giorni Mike Bongiorno, a pochi passi da uno dei quartieri più popolosi, che al tempo suscitava l'attenzione di pochi, ma dentro le cui mura si verificavano atrocità a danno di persone che avevano l'unica colpa di essere di un'altra religione, etnia, orientamento sessuale o di battersi per la propria libertà. Proprio quel *lager*, o meglio il suo perimetro murale, è stato oggetto recentemente di importanti interventi, che lo hanno reso un presidio di memoria e di educazione, come dovrebbero sorgerne tanti altri nel nostro Paese. Ancora ci tengo a ringraziare per la sua presenza il presidente Mattarella, che, insieme al Presidente della Repubblica austriaca, partecipò all'inaugurazione delle nuove installazioni, dando il senso di un popolo intero consapevole e maturo, di un'Italia che non vuole dimenticare. Combattere l'indifferenza è quindi, come eredi di coloro che hanno vissuto e subito quegli abomini, la nostra battaglia campale, perché è nell'indifferenza, a cui troppo spesso la nostra società cede, che l'odio trova il terreno fertile per germogliare. Per vincere questa battaglia è fondamentale - lo voglio dire con forza - ricordare il passato, ma agire con la stessa

auspicano la cancellazione di Israele, che - è bene ricordarlo - rappresenta un baluardo di democrazia e libertà imprescindibile *(Applausi)*, che ha dato una casa a coloro che hanno pagato il prezzo più alto dell'Olocausto. L'auspicio che voglio rivolgere in questa occasione, settantotto anni dopo la liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz, è che quello che diciamo oggi non resti un vuoto esercizio di retorica, ma possa diventare la realtà della nostra azione, sia qui dentro che fuori, nella nostra quotidianità. Solo con l'impegno costante di tutti potremo fare in modo di illuminare quel futuro che tanti giovani, come la piccola Anne, non hanno avuto l'opportunità di vivere.

ha detto parole amarissime, che credo abbiano colpito tutti noi e che costringono a porci interrogativi angosciati sul rapporto della nostra società con la memoria,

ma temo non priva di fondamento. Il rischio di una normalizzazione della Shoah e della sua derubricazione a fatto storico fra i tanti esiste davvero. Celebrare il Giorno della Memoria vuol dire proprio contrastare questa minaccia. La Shoah è stata una tragedia immane e unica non solo per le dimensioni dello sterminio, ma per le sue modalità tecnocratiche e burocratiche. Il progetto di eliminazione di un intero popolo fu pensato e praticato secondo una logica di pura efficienza industriale. Le vittime furono spogliate di ogni connotato umano e assimilate - come si compiacevano spesso di segnalare la propaganda e la pubblicistica nazionalsocialista - a un virus. Non era mai successo e non è successo nemmeno dopo, neppure in tragedie che, per ferocia e dimensioni, possono in qualche modo richiamare lo sterminio dei nazisti. Questa unicità della Shoah non va mai persa di vista. Al contrario, negli ultimi anni abbiamo assistito sempre più spesso a una banalizzazione della Shoah. Le accuse di nazismo e di genocidio sono state dispensate a cuor leggero, brandite a destra e a manca senza alcuna cognizione di causa; sono diventate quasi un luogo comune nel dibattito e nello scontro politico. Bisogna invece stare molto attenti, perché questa banalizzazione è esattamente l'anticamera dell'oblio. Non dobbiamo nasconderci il rischio, insito anche nello stesso Giorno della Memoria, di una ritualizzazione istituzionale del ricordo della Shoah, che può produrre esiti opposti a quelli per cui la giornata è stata istituita. I rituali diventano abitudini e l'abitudine spesso svuota di senso e di significato. Bisogna saper gestire invece la memoria, riconoscendo questo rischio e contrastandolo. Una via utile credo sia quella che indica spesso il capo rabbino di Roma Riccardo Di Segni, quando denuncia la tendenza a catalogare gli ebrei sterminati dai nazisti nell'anonima categoria di vittime. Per sentirle vive, per irrorare il ricordo del loro sterminio, quelle vittime vanno riconosciute per quello che erano prima di indossare il pigiama a righe, nella loro cultura distrutta dal nazismo, innanzitutto, e nella loro realtà. Forse parliamo troppo delle SS e troppo poco della ricchissima cultura ebraica che le SS di Hitler distrussero. Un discorso simile vale anche per i carnefici. La Shoah non ha riguardato solo chi accatastava i cadaveri nelle fosse comuni, ma anche tutti quelli che erano complici anche solo con il loro silenzio, quelli che guardavano facendo finta di non vedere, che si disinteressavano perché la faccenda non li riguardava, che chiudevano i porti agli esuli ebrei perché accoglierli avrebbe provocato troppi problemi e naturalmente quelli che erano invece complici attivi o che avevano varato le leggi razziali antisemite, come un'Italia che si è rapidamente assolta dalle proprie colpe e le ha troppo rapidamente rimosse. Sono lezioni che dovremmo tenere a mente non solo per quanto riguarda la memoria, ma anche per il loro buon uso nel presente, perché se è vero che vedere una Shoah dietro ogni angolo significa, nella sostanza, negare la Shoah, è anche vero che c'è una sua perversa e subdola eredità che permane. Ogni volta che affrontiamo un problema dimenticando che si ha a che fare con persone reali e vive e non con numeri, ogni volta che di fronte al razzismo o alle violazioni dei diritti umani ci rassegniamo o fingiamo di non vedere, è l'eco di quella lontana eredità che si fa sentire. A combatterla in ogni sia pur minimo suo elemento serve e deve servire la Giornata della Memoria.

al centro la foto in primo piano di Anne Frank giovane, sorridente e ancora ignara del suo tragico destino. Ricordo ancora ciò che provai mentre leggevo quelle pagine, un diario di vita familiare che perdeva precocemente la leggerezza che ti saresti aspettato da questo genere d'opera e assumeva velocemente la natura di una testimonianza straziante, facendoti comprendere il senso di impotenza e di stupore con il quale gli ebrei vissero il periodo che andò dall'introduzione delle leggi razziali fino alla deportazione, mentre intorno a loro gli altri, quelli che fino a poco tempo prima erano i colleghi di lavoro, i compagni di classe, gli amici d'infanzia, assistevano indifferenti allo sterminio. Nell'anno 2000, con la legge n. 211, l'Italia ha voluto riconoscere il 27 gennaio come Giornata della Memoria e di seguito anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione del 1° novembre 2005 ha designato la medesima data come Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Ma celebrare la Giornata della Memoria, come ha detto lei perfettamente, Presidente, come ci accingiamo a fare noi oggi e con le manifestazioni che domani si svolgeranno in tutta Italia, non è solo un adempimento formale, ma al contrario deve costituire l'occasione per scuotere le nostre coscienze e domandarci se stiamo facendo abbastanza se stiamo facendo abbastanza per contrastare i fenomeni di odio, di discriminazione, di violenza e di sopraffazione, se stiamo facendo abbastanza per ripagare con la nostra opera concreta il sacrificio patito dalle vittime della Shoah, se stiamo facendo abbastanza affinché ciò che è accaduto non si ripeta mai più. In questo senso, mi hanno molto colpito le parole della senatrice Liliana Segre, che ha dichiarato che oggi c'è quasi fastidio nel ricordare l'Olocausto e che di questo passo la Shoah finirà per essere appena un rigo nei libri di storia, così come sono rimasta colpita dalle parole dell'intervento della senatrice Segre la settimana scorsa in occasione della istituzione della Commissione straordinaria contro i fenomeni di discriminazione, violenza e odio, quando la senatrice ha rievocato i viaggi della memoria spesso vissuti dai visitatori con lo stato d'animo di una partecipazione a una gita ad Auschwitz, a metà strada tra una passerella dei potenti del mondo occidentale e una gita a una Disneyland della tortura contemporanea. La verità è che con il passare degli anni si dirada la possibilità di ascoltare i sopravvissuti e per questo la trasmissione della memoria dev'essere un atto ancora più rigoroso. D'altronde, la Giornata della Memoria non serve a far ricordare a chi non potrà più dimenticare ciò che è accaduto, ma serve a dire a chi è venuto dopo, a chi ha potuto godere dei fiori della pace e della democrazia, nati da queste macerie, quanto fragili siano le nostre libertà e quindi quanta cura e quanto impegno siano necessari per mantenerle vive. Ciò per evitare che qualcuno possa metterle in discussione o possa pensare di limitarle, a favore di un gruppo di persone e a discapito di un altro gruppo solo perché è percepito come diverso e quindi pericoloso. I superstiti della Shoah hanno vissuto la loro vita con l'insopportabile peso di dare forma e parole al male. Come ha scritto Rodolphe Gasché, la particolarità più terribile di Auschwitz fu il tentativo sistematico di impedire la formazione di storie e quindi di impedire ai posteri di poter narrare quell'orrore, di poter avere prove tangibili di ciò che era stato compiuto, di potere documentare la storia. Il peso della storia, della sua narrazione e della sua documentazione deve quindi gravare su di noi come un dovere morale da tramandare di padre in figlio, affinché nessuno possa permettersi di mettere in dubbio l'esistenza di ciò che è accaduto. Tutti dobbiamo avere ben chiaro che l'abisso della ragione è sempre pronto a generare i mostri dell'umanità, e nel farlo ne dobbiamo avvertire tutta la fatica: quella di coloro che si misurarono con gli abissi dell'orrore. Al tempo stesso, dobbiamo alimentare la fiamma della speranza, affinché non sia il ricordo rancoroso a guidare le nostre scelte, ma sempre la consapevolezza del bene, che sostiene i nostri passi e ci unisce in un ideale abbraccio a tutti coloro che, passando da un camino, sparirono nel vento ma sono ancora vivi nella nostra memoria. Questa Giornata è per loro che furono vittime; questa Giornata è per noi che dobbiamo ricordare affinché non accada mai più.

I ricordi possono sbiadire col tempo; la memoria, che oggi celebriamo, è invece un esercizio complesso e impegnativo, un compito che ci riguarda in prima persona, nessuno escluso. José Saramago ci ricordava che noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere, perché tenere viva la memoria è un atto di civiltà. Per questo il nostro Paese ha il dovere di educare alla memoria sin dalla scuola: proprio da lì, infatti, partì l'incubo delle leggi razziali, una delle pagine più dolorose della nostra storia. Nel settembre del 1938, il primo ad essere colpito dalla legislazione razziale fu il settore dell'istruzione, con l'esclusione degli ebrei dall'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado, dall'assistentato universitario e dal conseguimento della libera docenza; con l'esclusione dalle scuole di qualsiasi ordine e grado agli alunni ebrei. La scuola fu il punto di partenza e il centro della legislazione antiebraica, volto non solo ad escludere agli ebrei il percorso di formazione, ma a cancellarne le tracce anche da ogni strumento didattico. A farne le spese furono tanti docenti, tante bambine e tanti bambini, privati dell'istruzione e della conoscenza. Una di loro siede con noi tra i banchi del Senato e in quest'Aula abbiamo il privilegio di ascoltare la viva voce di chi è stato testimone dell'orrore nazifascista, di chi il coraggio della verità, di chi ha vissuto sulla propria pelle, su cui porta ancora i segni, il male incarnato. «I vuoti di oblio non esistono», scriveva E ancora: «Nessuna cosa umana può essere cancellata completamente e al mondo c'è troppa gente perchè certi fatti non si risappiano: qualcuno resterà sempre in vita per raccontare. E perciò nulla può mai essere praticamente inutile, almeno non a lunga scadenza». Le parole della Arendt sono un monito a non arrenderci, uno stimolo a portare avanti la memoria. Il nostro compito di legislatori è dunque permettere che la memoria di Liliana Segre, e con lei quella di tutti i testimoni della Shoah, resti viva. Quelle testimonianze hanno la capacità di formare gli anticorpi contro l'indifferenza, che saranno tanto più resistenti quanto prima si inizierà a raccontare. È dalla scuola che deve ripartire quel faticoso esercizio della conoscenza; è alla scuola e all'educazione che dobbiamo guardare se vogliamo che la memoria non sia solo la celebrazione di una giornata e che il male del passato si trasformi nell'urgenza del futuro. Primo Levi ci ricordava: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre». Non possiamo permetterlo. Sappiamo che il miglior strumento di conoscenza è l'esperienza diretta, come quello che fanno i nostri ragazzi durante i viaggi della memoria. Da consigliera della Provincia di Torino ho avuto la fortuna di accompagnare gli studenti delle scuole superiori ad Auschwitz e Birkenau, quello che il presidente Mattarella ha definito «la costruzione più disumana mai concepita dall'uomo. Uomini contro l'umanità». È il non luogo, l'inaudito, il mai visto, l'inimmaginabile. Fu un viaggio nella vertigine generata dal mare, in un baratro che si apre sotto lo sguardo. Dopo quell'esperienza nulla può essere come prima, i ricordi non possono più scolorire e le parole di Primo Levi diventano immediatamente lo stimolo alla memoria, come l'antidoto al male. Quei viaggi sono l'esempio di come la scuola sia educazione e conoscenza, di come l'uguaglianza, la libertà, la democrazia, il diritto e la pace si devono perseguire ogni giorno per non ricadere nel baratro. Sono il buon esempio di come la scuola possa formare oggi i cittadini di domani. *(Applausi)*.

perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre»: ha citato Primo Levi anche la mia collega Fregolent. Sono trascorsi settantotto anni da quel 27 gennaio del 1945, quando l'Armata rossa liberava Auschwitz, svelando al mondo le atrocità del campo di sterminio. Tutto intorno c'erano solo macerie, macerie morali e materiali, la devastazione della guerra, la privazione della libertà, il rifiuto e l'annientamento dell'identità degli esseri umani, la cancellazione di nomi, storie, famiglie e comunità, l'innocenza perduta per sempre, l'asservimento e l'umiliazione, l'assenza di forza e di capacità persino per piangere; la passività di tanti, troppi testimoni, l'abisso della viltà, il bene e il male. Sfogli le pagine del grande volume del Secolo breve e restano stampati capitoli intrisi di dolore, la fitta trama di un uso folle e disumano dell'ideologia, che ha portato a considerare i propri simili non uomini. La concezione più disumana mai concepita, «uomini contro l'umanità» disse il presidente Mattarella alcuni anni fa al Quirinale. C'è stato un tempo in cui dimenticare era più importante che ricordare. Troppo dolore, troppa sofferenza rendevano quel peso della storia insostenibile per chiunque, ma il ricordo infrange ogni tabù, sfida il tempo, l'orrore, l'angoscia e la sopraffazione. Si proietta verso il futuro, si tramanda alle nuove generazioni. Il ricordo genera gli anticorpi per l'indifferenza, una parola che certamente, non a caso, la senatrice Liliana Segre ha voluto fosse scolpita all'ingresso del memoriale della Shoah di Milano. Non c'è e non può esserci spazio per il sonno della memoria, non può esserci spazio per l'oblio, nemmeno quando il tempo inesorabile spegne a poco a poco la voce dei testimoni. La memoria lavora, come una goccia che scava la pietra, anche se può scivolarle sopra senza lasciare tracce. È una strana, ibrida divinità, avverte Barbara Spinelli, promette e minaccia al tempo stesso, risveglia le coscienze, ma una falsa memoria può anche renderle più ottuse, immobilizzarle. Mnemosine, la dea greca della memoria, ci obbliga precisamente a questo: a guardare dentro noi stessi, a studiare il passato che dorme o ci tormenta, che si camuffa o s'accampa davanti ai nostri occhi per schiarirci la via che stiamo percorrendo. un'odissea dell'Europa tra guerra e pace, alla fine giunse una non più sperata primavera di libertà. Ha vinto la vita, ha vinto la democrazia. Certo la memoria da sola non basta, non è sufficiente rievocare se poi non riusciamo ad offrire solide fondamenta alla definizione di un nuovo umanesimo europeo. Noi però non stanchiamoci mai di leggere le storie, di ascoltare le voci dei testimoni che hanno avuto coscienza della crudeltà dell'uomo, perché ci fortificano il cuore, illuminano il nostro presente e ci rafforzano nella determinazione a proseguire lungo il cammino della pace, oggi più che mai. *(Applausi)*.

per ricordare le vittime dell'Olocausto partendo da un giorno particolare, un giorno speciale, il giorno in cui si sono aperti i cancelli di Auschwitz e abbiamo avuto l'opportunità di riconciliare il genere umano con se stesso. È per questa riconciliazione che dobbiamo ricordare, come stiamo ribadendo tutti, anche la collega che mi ha preceduto. Dobbiamo avere memoria di quell'orrore. Dobbiamo rivedere e risentire insieme l'abisso. Dobbiamo ricordare quell'inferno per riconoscere, nel passato, che cosa inferno non è e dargli spazio e proteggerlo. Un passato che non ci sconvolge è un passato che non ci cambia, perché ricordare il passato trasforma il presente. Signor Presidente, se me lo concede, oggi vorrei soffermarmi, nei pochi minuti che ho a disposizione, proprio ed esclusivamente sul valore della memoria, ma non come contenitore di un tempo passato, un contenitore sicuramente prezioso, che va custodito e tramandato. Vorrei, invece, pensare alla memoria come ad un vaso di Pandora, che si svuota, si apre, sconvolge e stravolge tutto e quindi, cambia ogni cosa e ci ricorda di che sostanza siamo fatti o di che sostanza possiamo scegliere ogni giorno di essere o di diventare. Per farlo, chiaramente, non potrò usare le parole mie. Ho parole limitate e quindi prenderò liberamente in prestito le parole di Massimo Recalcati. Dobbiamo, colleghi e colleghe, considerare che il passato non è un corpo morto che giace; non è solo qualcosa che è accaduto e che va ricordato. Non è solo una commemorazione delle reliquie, ma il passato deve essere luce viva della trasformazione di quei sacrifici e di quell'orrore in qualcosa che liberi il presente, che ci trasformi, che ci riconcepisca.

Dalla memoria noi possiamo prendere tutto o solo un particolare. Io oggi voglio recuperare solo un particolare, un episodio, che Liliana Segre spesso racconta, di quando, nel campo di concentramento, ebbe l'opportunità, quasi l'occasione, di raccogliere una pistola da terra. Era lì e l'istinto forse la stava portando a raccogliere quella pistola. Era nell'abisso, era nell'inferno, era una giovane Liliana, impaurita, arrabbiata, che probabilmente aveva l'occasione di vendicarsi. In quell'abisso, Liliana Segre ha scelto di che sostanza voleva essere. Ha scelto a quale genere umano appartenere. Ecco la lezione della memoria: avere consapevolezza oggi che, anche nell'abisso, anche nell'inferno, si può sempre ancora scegliere di che sostanza essere. essere. Colleghi, non è vero che quando ci tolgono tutto alla fine non resta niente, perché, alla fine, rimaniamo sempre noi e possiamo scegliere di che sostanza essere.

Signor Presidente, settantotto anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz ha svelato al mondo l'orrore dello sterminio ebraico. Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi, perché quel male inferto a donne, uomini e bambini senza colpa è universale e non dovrà mai essere dimenticato. «Racconta, non ci crederanno, ma tu racconta e sopravvivi. Racconta per noi». È la fine di marzo del 1945 e una giovanissima Edith Bruck non ancora quattordicenne, arrivata in campo di concentramento dopo una marcia disumana, per poter avere una ciotola di zuppa è costretta a trasportare i cadaveri dei compagni nella tenda della morte

ci onora di essere seduta qui tra noi come senatrice a vita e che noi ringraziamo, missione di instancabile donna che racconta la sua storia. Questa commemorazione non deve essere però un esercizio retorico per rendere omaggio oggi a quel 27 gennaio del 1945 che ha segnato una delle pagine più tristi e più buie della storia dell'umanità. Il ricordo è l'unica via per vincere il buio dell'indifferenza. Solo la memoria può renderci davvero consapevoli del passato e del futuro che vogliamo. Conoscere la storia non basta. È necessario comprenderla, capirla e sentirla nella sua terrificante realtà perché - come ci ha insegnato Primo Levi - se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Solo così il ricordo di ciò che è stato diventa ispirazione per vincere l'indifferenza, per non voltarsi mai dall'altra parte, per battersi sempre e comunque in difesa del bene supremo della vita e della dignità umana. La libertà, la democrazia e l'uguaglianza sono il lascito che la Shoah ci ha affidato, sono un'eredità che va coltivata ogni giorno, lottando con le tante insidie esistenti, costruendo solidi antidoti contro i germi della discriminazione, della violenza e della sopraffazione. Memoria significa, allora, non solo prendere un'ulteriore coscienza su tutto ciò che avviene nel mondo a tutt'oggi, ma anche farne tesoro e declinare la comunità in termini di libertà, di uguaglianza e di rispetto dei diritti fondamentali. Da qui l'importanza dello studio della storia, la necessità di capire il Novecento, la necessità nelle nostre scuole di una didattica della memoria, di una nuova didattica della Shoah e dell'Olocausto, affinché si costruisca sin dalle aule scolastiche una coscienza civile condivisa e duratura, in cui tutti devono riconoscersi e che determini la formazione di cittadini consapevoli che si sentano parte di uno stesso destino. Permettetemi di ricordare ancora una volta oggi la legge approvata qualche giorno fa

per ottenere più risorse per permettere al maggior numero possibile di studenti di compiere un viaggio della memoria. È un'esperienza forte, fortissima, alla quale gli studenti devono essere adeguatamente preparati affinché possano trarne un vero insegnamento. Ma è certamente ciò che permette

sia emerso quanto le parole di Liliana Segre abbiano colpito tutti noi. Mi riferisco alle parole, più volte qui citate, sul fatto che la Shoah possa ridursi - è la preoccupazione che la senatrice evidenziava - tra qualche anno solo a un paio di righe a un rigo solo sui libri di storia. Perché queste parole forti ci hanno preoccupato e perché penso che sia importante che la politica se ne preoccupi? Penso che Penso che la politica debba chiedersi se possa esserci una tale eventualità, se davvero si possa immaginare che tutto ciò che è stato possa scomparire o essere semplicemente relegato a una parentesi. Penso che la politica si debba porre la questione di che cosa significhi fare memoria. Fare memoria - lo viviamo tutti noi, sempre - non è un esercizio semplice, perché significa andare ripescare cose che sono state sepolte. Spesso la memoria non è continuativa, ma è appunto un esercizio, per cui si deve procedere all'interno, scavare, recuperare, tenere insieme, costruire un legame. Ciò avviene in qualsiasi passaggio

si legge soprattutto all'ultimo anno delle scuole superiori e che viene ricordata soprattutto in questi giorni: mi riferisco a "Se questo è un uomo", di Primo Levi. Non mi soffermo sulla poesia che apre quel romanzo, ma mi soffermo su un grande esercizio di memoria che Primo Levi ci lascia, all'interno di quell'opera, in uno dei capitoli, che si intitola "Il canto di Ulisse". Signor Presidente, tutta l'opera è pensata come un viaggio all'inferno. Primo Levi sapeva che quello era l'inferno sulla terra e ben poteva ricordarlo. Egli ci racconta dunque, in quel capitolo, una vicenda particolare: aveva un'ora di tempo per andare a prendere il rancio e distribuirlo, insieme a un compagno, che era francese - si chiamava Jean e veniva chiamato "Pikolo" - e che voleva imparare l'italiano. A Primo Levi viene l'idea folle - dice lui - come folle era stato il volo di Ulisse, di spiegare l'italiano traducendo la Divina Commedia. Pensa dunque al canto di Ulisse e prova, facendo uno sforzo incredibile per far rivivere quei versi. Cerca di tradurli e fa fatica, perché la stanchezza, le difficoltà, il mondo in cui stava vivendo gli impediscono un esercizio facile. Egli però è tenace, scava dentro di sé, li cerca e fa in modo che quei endecasillabi escano. Prova a tradurli e fatica, fino

di un protagonismo, e cioè dell'esserci, dell'essere umano nell'ambiente, in quel mondo che aveva annullato l'umanità, che aveva provato l'annullamento dell'umanità, che aveva disumanizzato. Così, con forza, traduce quel «ma misi me» e sente che è vivo, si sente in vita e ci lascia questo esercizio di memoria e di vita nella memoria. Signor Presidente, far riemergere la memoria dice a noi, che persone vogliamo essere, il fatto di voler riscoprire la nostra umanità, cosa significa essere umani. La poesia aveva obbligato Primo Levi a scoprirsi nuovamente uomo e gli aveva dato una speranza. In quell'esercizio della memoria c'era una vittoria contro tutta la morte.

possa trasformarsi in futuro in qualche riga di storia ed essere abbandonata, la politica deve essere conseguente nel suo esercizio di fare memoria. E dovrebbe ricordarlo sempre; dovremmo ricordarlo tutti, ogni volta che esercitiamo il nostro ruolo di legislatori. Dobbiamo essere conseguenti e dobbiamo fare in modo di ricordare sempre che siamo ciò che siamo stati e che, nelle nostre scelte legislative, non possiamo dimenticare ciò che è stato.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, illustri ospiti presenti, quando si parla di Shoah, e cioè di quella tempesta devastante - questo vuol dire la parola che è stata costituita dallo sterminio del popolo ebraico sotto il regime nazionalsocialista in Germania e in altri Stati europei - si usa spesso l'espressione «mai più». Ci sono stati molti altri genocidi o tentativi di genocidio nella storia e molti altri gravi episodi di massacri di ebrei. Ma le dimensioni della Shoah, i milioni e milioni di vittime, il suo contesto moderno, con al centro il colto popolo tedesco, la sua programmazione industriale, il coinvolgimento di altre Nazioni di lunghissima civiltà come l'Italia, l'antichità plurimillenaria del popolo ebraico e la sua straordinaria influenza sulla civiltà europea e occidentale, lo rendono un fatto unico: un abisso di infamia, la negazione di ciò che è l'umanità. Giusto e doveroso dire mai più, e ricordare quanto avvenne, coltivarne la memoria, ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti, come la nostra cara collega Liliana Segre - oggi impegnata in altre commemorazioni e studiare quei fatti in tutti i loro aspetti. Tanto più che oggi c'è chi nega la realtà dello sterminio, e negare è premessa per replicare. Per questo il Parlamento italiano ha approvato nel 2016 una norma che fa del negazionismo della Shoah un'aggravante per chi compie o istiga a compiere reati. sulla base di esso. Non dobbiamo dimenticare che nella stessa Aula, dove pochi anni fa approvata questa legge e nel 2000 fu approvata l'istituzione del Giorno della memoria, nel 1938 furono approvate le infami leggi razziali. Conseguenza di quelle leggi - sia pure indiretta - fu, dopo pochi anni, la deportazione da Roma e da tutta Italia di migliaia e migliaia di ebrei, tra i quali il nonno della senatrice Mieli, che ci onora di essere nel nostro Gruppo. Pochissimi di loro fecero ritorno dai campi di sterminio. Non va dimenticato che a preparare quelle leggi ci fu il manifesto della razza, firmato solo da scienziati, tutti prestigiosi docenti universitari; scienziati di una scienza prona a un'ideologia, il cui antisemitismo aveva radici nei vari filoni dell'antisemitismo storico, tra cui, sia pure secondariamente, la radice cristiana, fatto che da cristiano è doloroso, ma doveroso ricordare. Ma in quell'ideologia era soprattutto forte l'aspetto "pretesamente" scientifico e ateistico, per il quale la selezione darwiniana era non solo la causa unica della nascita della specie umana, ma anche un valore sociale e politico. E, poiché le moderne comodità e l'idea - ritenuta inaccettabile - che ogni vita umana è degna avevano fortemente indebolito la selezione naturale, occorreva l'eugenetica e la soppressione di chi non era adatto e indeboliva la razza. Queste teorie, già allora assai diffuse, oggi non sono scomparse. Non dobbiamo poi dimenticare che, con la fondazione dello Stato di Israele, è arrivato l'antisemitismo vestito da antisionismo, a forte componente islamica, ma non solo. Ricordiamo - per limitarci ai fatti avvenuti in Italia - gli attentati a Fiumicino nel 1973 e, dodici anni dopo, con 48 morti e decine di feriti, e solo a pochi passi da qui, davanti alla grande sinagoga, l'attentato in cui morì Stefano Gaj Taché di due anni, e 40 furono i feriti, tra cui il fratello di Stefano. Ricordiamo anche le innumerevoli risoluzioni presso le Nazioni Unite contro lo Stato di Israele, più numerose di tutte le altre risoluzioni contro altre violazioni violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani sommate insieme. Dunque, mai più tutto questo. Mai più ritenere che ci sia chi non è degno di vivere e che lo Stato possa sopprimere il senso di umanità e le libertà naturali in nome di ideali o di esigenze più alte. Oltre alla memoria, oggi abbiamo un altro grande scudo, la Costituzione, che stabilisce principi e limiti invalicabili anche per le leggi stesse. In nessun modo potrebbero essere accettate e approvate norme come quelle del 1938, con le loro tragiche conseguenze, anche perché la libertà di espressione consentirebbe di opporvisi. La Costituzione va dunque difesa ogni giorno, mai disapplicata o interpretata in modo creativo e arbitrario. mai più dignità umana calpestata. Teniamo vivo il ricordo e voglio farlo ricordando il versetto di Isaia da cui è tratto il nome del memoriale della Shoah che c'è a Gerusalemme, lo Yad Vashem,

Signor Presidente, con riferimento alla questione posta dal senatore Potenti, si rappresenta quanto segue. La marmettola è un prodotto dell'estrazione della lavorazione del marmo e si presenta sotto forma di fango. Quest'ultimo è sottoposto a disidratazione e recupero delle acque, e successivamente stoccato per essere gestito come rifiuto, pertanto soggetto o a smaltimento oppure al recupero. Ciò permesso, si precisa che la competenza in ordine al controllo degli impianti, e più in particolare sulla corretta gestione dei rifiuti, spetta agli enti territoriali. Va sottolineato comunque che se, come nel caso dell'interrogazione, la marmettola finisce nei corpi idrici, si genera il fenomeno della copertura del substrato naturale dei fiumi da sedimenti con conseguente aumento di torbidità delle acque e ripercussioni sull'ambiente fluviale interessato. Per quanto concerne le vicende che riguardano la società Venator rammentate dall'interrogante, la Regione Toscana informa che ha avviato da oltre un anno un confronto con la società per affrontare la necessità di messa a deposito di importanti quantità di gessi rossi, atteso che oggetto del confronto è anche la riduzione di produzione del rifiuto mediante modifiche ai cicli produttivi, che comporterà a regime una minore necessità di scarti del settore del marmo. Inoltre, allo stato attuale non sono in essere atti limitativi alla produzione da parte della Venator né a qualsiasi forma di conferimento, per quanto è noto che la disponibilità di volumetrie presso la ex cava di Montioni è in esaurimento. La Venator ha altresì ricevuto la concessione per l'autorizzazione di un impianto di stabilizzazione del fango per l'ottenimento di materiali *end of waste*, oltre ad aver disposto la presentazione di una valutazione di impatto ambientale per un progetto di ripristino. Infine, la Regione Toscana specifica che non risultano istanze inevase da parte dei produttori del rifiuto in argomento per l'autorizzazione al deposito temporaneo. Riguardo alla valutazione degli effetti della marmettola nei corsi d'acqua delle Province di Massa Carrara e Lucca, si rappresenta che dal 2017 al 2019 è stato realizzato il progetto Cave a seguito di deliberazione regionale n. 945 del 2016, avente il principale principale obiettivo di migliorare la gestione ambientale delle cave attraverso l'attività di controllo e la realizzazione di studi e ricerche, grazie allo stanziamento di risorse umane e strumentali dedicate. Dalle attività di suddetto progetto è emerso che le situazioni più critiche si osservano nel fiume Frigido e nel torrente Carrione (bacino Toscana Nord), dove è visibile il fenomeno della copertura prima descritto, sia come depositi e sia con episodi di aumentata torbidità delle acque. Se gli effetti sulla qualità ecologica dell'ambiente fluviale sono evidenti, va precisato che le condizioni sui due corsi d'acqua sono leggermente migliorate rispetto a quando veniva praticato abitualmente lo scarico della marmettola dalle segherie di marmo prossime ai corsi idrici. Inoltre, dal secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque 2021-2027 del distretto dell'Appennino settentrionale, emerge che lo stato ecologico del torrente Carrione, suddiviso nei corpi idrici torrente Carrione monte e torrente Carrione valle, risulta rispettivamente scarso e sufficiente. Per entrambi i corpi idrici, lo stato chimico risulta essere non buono. Parallelamente, allo stato ecologico del fiume Frigido, suddiviso nei corpi idrici fiume Frigido-canale Secco-Alberghi monte e fiume Frigido-canale Secco-Alberghi a valle, risulta rispettivamente buono e sufficiente. Lo stato chimico corrisponde a buono nel primo corpo idrico e non buono nel secondo. In questo caso, c'è stato un miglioramento sia dello stato ecologico che dello stato chimico nel corpo idrico fiume Frigido-Alberghi monte, rispetto ai risultati del precedente aggiornamento del piano di gestione delle acque. Infine, la Regione Toscana segnale che il 28 novembre scorso è stato convocato dalle Province di Massa Carrara e Lucca un tavolo di confronto, a cui erano presenti i rappresentanti delle categorie economiche sociali del settore, con l'intento di elaborare e inviare alla Regione proposte finalizzate al superamento delle criticità contingenti. Nel rammentare che, a tutela dei corpi idrici è possibile prescrivere a tutte le cave l'adozione di accorgimenti relativi alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento anche attraverso l'applicazione di quanto prescritto nella legge regionale n. 20 del 2006 e il relativo regolamento di attuazione, questo Ministero nell'ambito delle proprie prerogative continuerà nelle dovute interlocuzioni con le amministrazioni interessate.

causa di un richiamo che il Ministero all'epoca volle fare alla Regione Toscana per incentivare iniziative migliorative. Allo stesso tempo la ringrazio di aver ricordato lo stato della situazione amministrativa, che vede Regione Toscana e società Venator impegnate a tentare di risolvere la questione del ricovero dei residui della lavorazione successiva all'estrazione del biossido di titanio. Mi conforta il fatto che ci sia una regolarità delle situazioni amministrative, che permetteranno certamente all'azienda di studiare soluzioni migliorative verso quella pratica chiamata *end of waste*, che è una delle soluzioni assolutamente auspicabili, vista anche la quantità dei materiali che fino ad oggi sono stati ricoverati nella discarica

sull'ambiente, quando in realtà sappiamo che spesso il ritardo nell'azione amministrativa - lei lo ha ricordato, quando ha rammentato le competenze degli enti locali

Quindi, anche a nome del mondo produttivo, che con questa interrogazione ho inteso ricordare, la ringrazio per la risposta

sicuramente, dopo le esperienze passate, rispondere a questa emergenza.

Signor Presidente, con le interrogazioni in oggetto, focalizzate in particolare sul verificarsi di un evento suicidario all'interno della casa circondariale di Torino e, più in generale, sull'aumento dei suicidi dei detenuti all'interno degli istituti di pena del Paese, si avanzano quesiti in ordine all'assunzione di iniziative finalizzate ad arginare il fenomeno nonché a ridurre il sovraffollamento. Orbene, come evidenziato in sede di risposta ad interrogazione di pressoché analogo tenore, si assicura che l'attenzione al tema dei suicidi in carcere è massima e continuo sarà l'impegno che sarà profuso dall'amministrazione a mezzo del preposto Per dovere di precisione, si riporta la sequenza storica, dal 2009 ad oggi, del numero dei suicidi: 59 nel 2009, 63 nel 2010 e nel 2011, 57 nel 2012, 42 nel 2013, 43 nel 2014, 39 nel 2015 e nel 2016, 48 nel 2017, 62 nel 2018, 53 nel 2019, 62 nel 2020, 57 nel 2021 e 84 nel 2022, nel 2022, sino al 16 gennaio 2023. Certamente, siffatti numeri non possono che destare impressione e spingere all'individuazione e alla messa in opera di doverose soluzioni che, come si vede, affondano le radici

risultano emanate varie circolari, tra cui citerò le più significative negli ultimi vent'anni, come quella emanata in data 12 maggio 2000, recante: "Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario: linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri";

Nell'ultimo decennio, inoltre, tale attenzione si è maggiormente consolidata ed è stata condivisa con l'amministrazione della Salute, tanto che il 19 gennaio 2012, in seno alla Conferenza unificata Stato-Regioni, è stato sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" e nel 2017 è stato sottoscritto il "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti", con lo scopo di fornire linee guida ai livelli regionali al fine di consentire la successiva redazione dei protocolli locali, con la più ampia condivisione e concretezza tra le parti, sanitaria e penitenziaria. 11 ottobre 2017, sono state divulgate ai provveditorati regionali e a tutte le direzioni degli istituti penitenziari le indicazioni fomite dall'Accordo della Conferenza unificata del 27 luglio 2017, con il quale, sinteticamente, viene dato impulso a una fattiva collaborazione tra il DAP e le aziende sanitarie territorialmente competenti, al fine di creare i presupposti per alleviare, in via preventiva, l'eventuale disagio sofferto dalla persona privata della libertà personale e, in secondo luogo, delineare ambiti di intervento. È stato promosso il congiunto impegno di tutte le figure professionali che operano all'interno degli istituti penitenziari. nell'accordo vengono previsti, tra l'altro, il modello di lavoro interdisciplinare e la presa in carico congiunta, attraverso cui si sviluppa una collaborazione sinergica tra le varie figure professionali coinvolte, con l'obiettivo di lenire il disagio della persona offrendo vicinanza e supporto sociale. Successivamente, i concetti di cui sopra sono stati altresì ribaditi con la circolare del 3 maggio 2019, recante: "Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico". merita menzionare la recente nota del 2 luglio 2020 a firma del direttore generale dei detenuti e del trattamento, con la quale si raccomanda massima prudenza e attenzione nella percezione di possibili segni di disagio psichico o comunque di alterazione comportamentale dei ristretti, prevedendo un'assistenza psicologica più ampia. Inoltre, in considerazione dell'aumento dei decessi e dei suicidi nel corrente anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori d'istituto del territorio nazionale, il DAP, con nota circolare dell'8 agosto 2022, n. 3695/6145 (precisando che l'interrogante troverà i dati meglio specificati nel documento scritto), ha ribadito a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate, in particolare dal 2016 in poi, rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute, avviando sollecitamente un percorso nazionale di "intervento continuo" sul tema, attraverso il quale il dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari, siano tutti coinvolti, in una prospettiva di rete, nella prevenzione di tali drammatici eventi (nota dell'8 agosto 2022). In particolare, è stato chiesto ai provveditori regionali di verificare se, nei distretti di competenza, siano stati stipulati i Piani regionali di prevenzione. E ciò, ove gli stessi manchino, al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso l'interlocuzione con le rispettive autorità sanitarie. l'importanza del ruolo fondamentale all'uopo svolto dallo *staff* multidisciplinare, evidenziando la necessità che agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si sono manifestati un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui cosiddetti casi silenti, riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare. Su questo versante, dunque, è necessario che ogni direzione, unitamente ai componenti dello *staff*, abbia un'adeguata strategia per intercettare i soggetti che rischiano di rimanere invisibili. Sono stati definiti, altresì, gli ambiti potenzialmente critici verso i quali tutti gli operatori addetti alla gestione della persona detenuta devono essere adeguatamente indirizzati per cogliere eventuali segnali di pericolo (ingresso e accoglienza, colloqui con i familiari, flusso di corrispondenza, fasi pre e postprocessuali, comunicazioni di eventi traumatici, comportamenti anomali, tendenza all'isolamento, prossima dismissione e così via). È stata evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con l'ordine degli avvocati, al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto nel caso emergano situazioni di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti, nonché a livello locale con la magistratura e i garanti. È stata sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso, che tenga conto essenzialmente dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei *peer supporter*, modalità chiusura della procedura. Inoltre, in un'ottica di oculata gestione complessiva delle situazioni di disagio delle persone detenute, è necessario che particolare attenzione sia riservata al momento delle assegnazioni definitive in istituto e alle richieste di trasferimento, privilegiando le strutture penitenziarie che, per l'adeguata offerta sanitaria e trattamentale, siano in grado di soddisfare meglio le esigenze di presa in carico delle problematiche di disagio personale dei soggetti ristretti. Da ultimo, è stata sollecitata l'attivazione di giornate di studio e confronto collettivo sul tema della prevenzione suicidaria a tutti i livelli dell'organizzazione, onde favorire un coinvolgimento il più possibile esteso e la partecipazione del personale dell'area sanitaria in servizio negli istituti. Onde monitorare la presenza degli indicati piani regionali e la successiva sottoscrizione di piani locali, l'amministrazione ha provveduto a implementare le funzionalità dell'apposito applicativo informatico. Per completezza, si evidenzia che il *budget* relativo al capitolo

articolo 80 OP all'interno degli istituti di pena e, in special modo, di dare attuazione alle vigenti direttive concernenti la prevenzione delle condotte suicidarie delle persone detenute. Tali risorse, che si aggiungono a quelle già assegnate per il corrente anno nei mesi scorsi, sono state ripartite tra i provveditorati regionali, con l'invito rivolto a questi ultimi di procedere alla successiva ripartizione tra gli istituti del distretto di competenza, impegnando tutti i fondi disponibili, elevando sino al limite delle 64 vacazioni orarie le convenzioni già stipulate per un numero inferiore, stipulando nuove convenzioni con i professionisti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 132 del regolamento di esecuzione. Con riguardo all'annoso problema del sovraffollamento, non secondario, dei diritti dell'uomo (CEDU) Torreggiani del 2013, allo scopo di arginare il fenomeno, si è proceduto con l'individuazione, nell'ambito delle disponibilità esistenti, di spazi immediatamente utilizzabili e contemporaneamente sono stati progettati nuovi istituti. Nel tempo quindi, già dal marzo sono stati istituiti ufficialmente l'Applicativo spazi/detenuti (ASD) e relativo gruppo di lavoro, con il quale sono state fornite ulteriori indicazioni riguardanti l'allocazione degli spazi vitali minimi, stabiliti dalla Corte europea, diventando questo strumento informatico, allo stato, il sistema più avanzato per definire l'insieme di relazione tra detenuti e spazi detentivi. Tale applicazione consente non soltanto di conoscere il numero dei detenuti presenti nei singoli istituti, ma anche la loro corretta collocazione all'interno di ogni istituto (camere di pernottamento) e lo spazio disponibile per ciascun individuo, consentendo così di verificare in tempo pressoché reale il rispetto dei parametri CEDU e le eventuali violazioni, con conseguente ripristino della legalità. Detto applicativo è ben utilizzabile altresì dalla magistratura di sorveglianza, preposta per legge alla vigilanza sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. presso le carceri nazionali risulta un totale di 56.178 persone, di cui 55.702 effettivamente presenti in istituto, rispetto a una capienza pari a 51.340 posti, di cui 3.696 non disponibili a vario titolo, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 117,69 per cento. La competente direzione generale, laddove necessario, dispone provvedimenti deflattivi delle sedi penitenziarie che presentano un maggior indice di sovraffollamento. Occorre precisare che lo stato d'emergenza legato alla pandemia ha determinato, nel biennio 2020-2021, un congelamento dei provvedimenti di sfollamento, con l'adozione di provvedimenti di trasferimento adottati soltanto per gravi motivi di sicurezza, di salute o di giustizia. In ogni caso, alla data odierna, dagli applicativi in uso risulta che nessun detenuto è allocato in violazione dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Riferito quanto sopra, si evidenzia che il DAP è attualmente impegnato in un programma teso all'aumento del numero dei posti detentivi, mediante il recupero di agibilità di quelli indisponibili per carenze manutentive, nonché all'edificazione di nuovi padiglioni penitenziari già attivi, come pure la riconversione a uso detentivo di strutture demaniali dismesse, in particolare caserme, aventi caratteristiche tali da poterne prefigurare, con prevalenti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, un possibile adattamento a istituto penitenziario. Tra il 2020 e i primi mesi del 2021, sono stati ultimati e attivati quattro nuovi padiglioni da 200 posti ciascuno, presso gli istituti di Parma, Trani, Lecce e Taranto. Attualmente, sono in fase di collaudo, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo padiglione da 92 posti, destinato all'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis*, presso la casa circondariale di Cagliari, e il padiglione da 200 posti, presso la casa di reclusione di Sulmona. Entro il 2023, inoltre, dovrebbero essere ultimati il padiglione da 200 posti che si sta realizzando presso la casa circondariale Bologna e quello da 400 posti in costruzione presso la casa circondariale di «Roma Rebibbia». Tra gli interventi avviati per il riadattamento e il riuso di strutture militari dismesse, si annota quello relativo alla caserma Rotilio Barbetti di Grosseto, imminente presa in consegna da parte dell'amministrazione penitenziaria, da riconvertire in istituto da 400 posti. Inoltre, effettuati i relativi appalti dei lavori, entro il 2025 dovrebbero essere ultimati il nuovo padiglione da 200 posti presso la casa circondariale di Bologna e il nuovo istituto di Forlì da 250 posti. nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, è stata inoltre prevista la realizzazione di nuovi otto padiglioni da 80 posti detentivi, da edificarsi in aree già nella disponibilità di quest'amministrazione, quali sedi di istituti di pena, di pena, a Vigevano, Rovigo, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara e Reggio Calabria Arghillà, con il duplice obiettivo sia di ampliare la recettività del sistema penitenziario nazionale, sia di favorire una permanenza nei luoghi di detenzione più dignitosa. Il *format* di tali padiglioni detentivi, ispirazione fortemente trattamentale, è stato elaborato dalla commissione per l'architettura penitenziaria, costituita nel gennaio 2021, e la concreta esecuzione di tali opere è stata affidata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui si è avviata un'opera di costante collaborazione, finalizzata alla tempestiva attuazione dei progetti. La realizzazione di tali otto padiglioni dovrà essere ultimata entro il 2026 e produrrà ulteriori 640 640 posti detentivi; ciò consentirà di contrastare con maggiore adeguatezza ed efficacia la problematica relativa alla condizione di sovraffollamento che affligge il sistema penitenziario, nonché di assicurare una maggiore disponibilità di spazi utili per il superamento dell'attuale criticità legata, anche e soprattutto, alla grave mancanza di superfici e ambienti per le attività trattamentali. Quanto all'evento critico questo si è verificato in data 10 novembre scorso, allorquando, in base alle attuali informazioni acquisite, la polizia penitenziaria locale si avvedeva che il detenuto R.A. aveva compiuto un gesto anticonservativo mediante impiccamento. Naturalmente, venivano avvisati tempestivamente la sorveglianza generale, il medico, l'infermiere e gli operatori del 118, peraltro già presenti in istituto. Purtroppo, i tentativi di salvare il detenuto risultavano inutili e, alle ore 00,15 il medico ne dichiarava il decesso. Dell'evento venivano quindi informati il pubblico ministero di turno e uno degli avvocati del detenuto. Emerge inoltre che il signor R.A. non era alla prima esperienza detentiva e all'atto dell'ingresso non necessitava, secondo la valutazione del sanitario, di attenzione specifica. Quanto sopra precisato e ferme le valutazioni della preposta autorità giudiziaria, come usualmente avviene, è stata attivata apposita indagine ispettiva condotta dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, tesa ad accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'evento. Infine, in ordine all'adozione di misure alternative al carcere, allo stato si evidenzia il recente intervento normativo di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, contenente, appunto, tra le altre, la riforma delle pene sostitutive e delle pene detentive brevi. Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l'efficienza complessiva del processo e della giustizia penale. Si tratta infatti di pene diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di quelle detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale, con ciò realizzando un'anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione. L'entrata in vigore del complesso normativo sinora descritto, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata - come noto - differita, per effetto della previsione 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con la legge n. 199 del 2022, al 30 dicembre 2022, per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. Il differimento è stato pertanto contenuto entro la data indicata, trattandosi di un lasso di tempo ritenuto sufficiente al fine indicato e che permette, altresì, di mantenere gli impegni in relazione al PNNR. Merita infine segnalare gli interventi nello specifico settore disposti con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio Grazie

e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore; b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le Regioni; d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria». All'articolo 1, comma 858 si autorizza a bandire, nell'anno 2023, ed in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale; all'articolo 1, comma 864, si autorizza l'assunzione straordinaria di un del corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di 250 unità per l'anno 2023, 250

dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023. la rassegna di quanto è stato fatto, si sta facendo e si farà - nella prospettiva del miglioramento delle condizioni di vita e del livello di attenzione del Ministero su questi problemi - ho concluso.

direi - alle mie interrogazioni. Lo ringrazio anche per la comprovata cultura garantista di una vita che, naturalmente, mi ha fatto ascoltare le sue parole con particolare attenzione e con una certa apertura.

84 suicidi nelle nostre carceri lo scorso anno: è un numero altissimo; per intenderci, più o meno la metà delle persone morte in carcere sono morte per suicidio. A pensarci, è una statistica che fa fa inorridire, fa impressione. La ragione per la quale questi suicidi avvengono è che le nostre carceri hanno una serie di problemi enormi, alcuni dei

Spesso i suicidi avvengono nelle sezioni cosiddette dei nuovi giunti, dove le persone hanno la prima accoglienza, il primo *shock* e il primo trauma. però, è che non c'è soltanto un problema di tipo strutturale; ce n'è uno sicuramente di sovraffollamento, ma questo è dovuto al fatto che le carceri sono diventate il ricettacolo delle nostre marginalità.

legati agli stupefacenti, che sono anche una patologia, in un certo senso, quando si crea una dipendenza, e noi abbiamo una legislazione soprattutto punitiva per quel fenomeno.

Tutto questo crea una sorta di miscuglio e di *mix* micidiale, che naturalmente fa sì che le nostre carceri di fatto siano

peccato però che le cose che fate non siano sempre conseguenti, perché non posso dimenticare che la legge di bilancio, oltre alle assunzioni che lei ha ricordato, prevede 9,5 milioni di tagli al DAP; basta infatti parlare col direttore di una delle nostre carceri per sapere che è difficile anche mettere insieme il

come massimo della pena; un reato del tutto inutile e una pena stabilita soprattutto per garantire la possibilità delle intercettazioni, più che per la gravità del fatto, come spesso avviene. Si tratta quindi di una visione del diritto penale completamente distorta. Come dico spesso quando interloquisco col suo Ministero, signor Vice Ministro, noi ascoltiamo delle belle parole, coltiviamo una speranza che diventino realtà, però da opposizione devo dirle che il vostro comportamento e i fatti concludenti che abbiamo visto sinora vanno esattamente nella direzione contraria al risolvere i problemi della giustizia e in particolare questo della condizione carceraria, che è uno dei grandi scandali del nostro Paese.

Signor Presidente, ringrazio anche il senatore Scalfarotto per la garbata replica e rispondo volentieri all'interrogazione proposta dal senatore Giorgis. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti, riferito di eventi suicidiari occorsi in pochi mesi presso il carcere torinese ed evidenziata la tragica sequenza di suicidi

evidenziata la tragica sequenza di suicidi a livello nazionale, nonché le criticità esistenti in generale in tema di salute in carcere, in tema di scarsità del personale penitenziario ed in tema di criticità dello stato di manutenzione e ristrutturazione degli edifici penitenziari, hanno avanzato precipui quesiti in ordine alle iniziative che si intendano adottare e volte alla soluzione delle problematiche indicate. Poiché i quesiti posti risultano altresì avanzati in sede di interrogazione a risposta orale, è opportuno richiamare quanto già riferito in data 1° dicembre 2022 con le opportune precisazioni, anche a seguito della successiva esposizione delle linee programmatiche. Ciononostante, in via preliminare va ribadito come non si possa che restare sgomenti di fronte agli atti di suicidio che accadono nelle nostre carceri ed anche i quattro episodi di Torino confermano la gravità della situazione. Come già indicato in varie occasioni, ribadisco che l'amministrazione profonderà il massimo impegno (come ha cercato di fare) e attenzione alle politiche concernenti l'amministrazione penitenziaria, avendo ben a mente le gravose responsabilità che derivano dall'inderogabile dovere di dare corretta attuazione ai precetti scolpiti nell'articolo 27 della Costituzione. Si agirà quindi contestualmente sul piano relativo ai luoghi di esecuzione della pena e su quello relativo agli operatori penitenziali tutti, nonché naturalmente su quello relativo ai detenuti, per i quali lo Stato assume in carico il dovere di tutela degli incomprimibili diritti alla salute fisica e psichica e a un'esecuzione della pena degna e volta alla rieducazione (come previsto appunto dall'articolo 27), il tutto garantendo la sicurezza interna ed esterna agli istituti di pena. L'attenzione alla sanità penitenziaria dev'essere e sarà massima. Gli interventi saranno quindi rivolti alla tutela della salute, sia in generale, sia delle categorie fragili, quali i tossicodipendenti, i dipendenti in genere le persone con disagio psichico, risultando evidente la distanza da colmare prima di poter affermare l'effettività della tutela della salute nelle nostre carceri. Obiettivo primario perseguito è quello di individuare, possibilmente fin dall'ingresso, le persone con problematiche da dipendenza, con patologia psichiatrica o con rischio suicidario, per attivare immediate azioni di sostegno e promuovere i necessari interventi sanitari, sociali e psicologici. Va ovviamente implementato il coordinamento con le autorità sanitarie locali, con gli enti locali e con le comunità terapeutiche. Analoga attenzione dev'essere rivolta alla delicata tematica delle REMS, sulle quali, com'è noto, è intervenuta la Consulta, con decisione del 22 gennaio 2002. Dal punto di vista del personale, continuerà e sarà implementata, oltre alla doverosa e costante formazione, l'azione di incremento della dotazione organica, portando a termine altresì le procedure concorsuali già iniziate. L'implementazione riguarderà il personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria, quello del comparto funzioni centrali, con attenzione alle varie figure, posto che la carenza organica rappresenta una seria criticità in considerazione dei compiti e delle responsabilità loro attribuite, certamente fondamentali per il funzionamento degli istituti penitenziari e per l'opera di vigilanza e rieducazione dei condannati. In ordine agli istituti penitenziari, si continuerà sulla linea di interventi di innovazione e modernizzazione delle strutture penitenziarie, attraverso la costruzione di nuove carceri e di nuovi padiglioni, nonché attraverso l'ampliamento e l'ammodernamento delle attuali, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico. Ovviamente do per acquisiti tutti i dati che mi sono permesso prima di rappresentare e che sono già noti all'interrogante, per quanto già accaduto in seguito alle sollecitazioni mosse nei confronti del Ministero. Verranno altresì implementati sistemi di sorveglianza e controllo, anche attraverso un ammodernamento tecnologico degli apparati, con specifico riferimento alla videosorveglianza e a un sistema antidroni. Si interverrà poi in maniera incisiva per il miglioramento della qualità della vita del personale di Polizia penitenziaria, anche in termini di idoneità e vivibilità degli ambienti lavorativi. Quanto all'attuazione della recente riforma legislativa in materia di pene sostitutive di quelle detentive brevi, la relativa entrata in vigore è stata semplicemente differita - come noto al collega Giorgis - al 30 dicembre scorso, per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici, senza venir meno agli impegni assunti in relazione al PNRR. L'ambizioso programma indicato non può e non dev'essere intaccato dalle rimodulazioni delle previsioni di spesa previste nella legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, che non determineranno un ridimensionamento dei livelli essenziali dei servizi e della sicurezza nell'ambito degli istituti penitenziari, considerato che obiettivo del prossimo triennio sarà quello di riorganizzare e meglio efficientare tutti i servizi di istituto, in un quadro di ammodernamento delle strutture e degli impianti tecnologici anche destinati alla sicurezza, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale. sono finanziati con i fondi di parte capitale già iscritti in bilancio a legislazione vigente, inclusi gli stanziamenti autorizzati dal Fondo complementare al PNRR, e con le maggiori risorse per nuovi investimenti assegnate con la Sezione II della stessa legge di bilancio per il triennio 2023-2025. Per meglio chiarire, ad esempio, una significativa componente di risparmio è quella delle traduzioni dei detenuti per motivi di giustizia: l'implementazione, sempre con fondi di investimento, delle salette multi-video-conferenze all'interno degli istituti penitenziari ha consentito un considerevole abbattimento del numero delle traduzioni,

istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti: a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore; b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le Regioni; d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria». All'articolo 1, comma 858 si autorizza a bandire, nell'anno 2023, ed in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità

nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di 250 unità per l'anno 2023, 250 unità

per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

Con specifico riferimento al carcere di Torino, alla stessa data, risultano effettivamente presenti 1.370 detenuti, rispetto a una capienza regolamentare di cui 60 non disponibili, allo stato, a vario titolo, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 131,98 per cento. In ogni caso, dagli applicativi in uso risulta che nessun detenuto è allocato in violazione dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Passando ai singoli casi evidenziati dagli interroganti, dalle istruttorie sinora espletate risulta quanto segue. Il decesso del signor K.M.Z., di origine pakistana, si è verificato in data 24 luglio 2022, allorquando, in orario notturno, l'agente addetto alla vigilanza della sezione, mentre effettuava un giro di controllo, notava che il detenuto si era creato un cappio con un lembo di lenzuolo e si era legato alla finestra della camera di pernottamento. Venivano subito attivate le previste procedure di soccorso, provvedendo a tagliare la corda e a spostare il corpo del signor K.M.Z. per permettere le manovre di primo soccorso da parte del medico di turno. Veniva chiamato il 118 che, dopo aver eseguito il tracciato cardiaco, non poteva far altro che constatare il decesso del ristretto. Sono stati informati il magistrato di turno e le altre autorità competenti. Come usualmente avviene in queste situazioni, è stata attivata la prevista indagine ispettiva condotta dal Provveditorato regionale competente e volta ad accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'evento. 15 agosto 2022 presso la sezione Articolazione per la tutela della salute mentale (ATSM). In presenza dell'infermiere, la sorveglianza e il personale di Polizia penitenziaria presente faceva accesso nei locali di detenzione ove si appurava che il detenuto aveva il volto coperto da un sacchetto di plastica. Immediatamente, venivano avvisati la sorveglianza generale e il medico di guardia, che proseguiva le manovre rianimatorie iniziate dall'infermiere, ma senza successo. Dell'evento veniva informato per le vie brevi, tramite il cappellano, il padre del detenuto e se ne dava comunicazione anche al pubblico ministero di turno, il quale disponeva di trasportare la salma presso l'istituto di medicina legale di Torino a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'esame autoptico. Il 17 novembre 2022, il Provveditorato regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ha comunicato gli esiti dell'ispezione amministrativa condotta in relazione al decesso del detenuto G.A. e si è in attesa delle verifiche in ordine all'eventuale sussistenza di profili di responsabilità disciplinare a carico dei singoli operatori penitenziari. Il terzo evento suicidiario citato risulta occorso in data 28 ottobre e riguarda un cittadino di origine del Gambia. L'addetto alla vigilanza della sezione, con l'ausilio di altre unità di Polizia penitenziaria, ha provveduto dunque ad aprire la porta della camera di pernottamento, liberando il detenuto dal cappio e adagiandolo sul pavimento; il personale sanitario, nel frattempo accorso, ha iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite invano dal personale del 118 sopraggiunto. Anche in tal caso, è stata informata l'autorità giudiziaria e poi attivata la prevista indagine ispettiva, volta ad accertare cause, circostanze e modalità dell'evento, nonché a verificare se siano state attivate tutte le procedure operative volte a cogliere i possibili rischi suicidari. Infine, in data 10 novembre 2022 risulta verificatosi il quarto evento citato. Risultano effettuate le previste procedure di soccorso, avvisata la sorveglianza generale, il medico, l'infermiera e gli operatori del 118, i quali erano già presenti in istituto a causa di un malore occorso ad altro detenuto ubicato al secondo piano. Purtroppo, anche in questo caso, vani sono stati i tentativi di rianimazione. Dell'evento venivano informati il pubblico ministero di turno e uno degli avvocati del detenuto, affinché informasse i familiari. Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro della risposta. Devo dire che quattro suicidi in neanche un anno nella sola casa circondariale di Torino sono davvero qualcosa di drammatico e inaccettabile. Negli altri istituti penitenziari del territorio nazionale la situazione, purtroppo, non è meno preoccupante. Come ha ricordato anche il Vice Ministro, i morti per suicidio dall'inizio dell'anno sono oramai più di Queste morti rappresentano una sconfitta per le istituzioni e per l'intera società, perché il carcere, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione, dev'essere non solo l'*extrema ratio*, ma luogo di ricostruzione di opportunità, mai di morte.

mi chiedo quali siano gli interventi immediati e di medio periodo che il Governo intenda assumere. Si tratta di interventi che in alcuni casi non possono essere rinviati a un futuro indeterminato, ma devono muoversi su diversi piani: non c'è una risposta semplice che possa scongiurare il rischio che si consumino ulteriori morti in carcere, ma occorre agire su tanti aspetti. C'è il tema serissimo del sovraffollamento:

abbiamo istituti penitenziari che non sono in grado di adempiere a quella funzione garantendo che la pena sia opportunità di reinserimento e trattamento capace di offrire formazione,

da ciò che ho sentito in ordine alla scelta di procedere, per affrontare questo problema, nella sola direzione di costruire nuove carcere e nuovi padiglioni. Certo, il tema del sovraffollamento è urgente e da affrontare in maniera radicale, ma non è che lo si debba fare in un'unica direzione. Ho sentito numeri che prefigurano un piano di edilizia carceraria significativo, ma le chiedo: se imboccassimo anche la strada che pure il ministro Nordio pare aver detto di voler provare, cioè quella del carcere come *extrema ratio* e di un investimento sulle misure alternative, perché si si prefigura questa sola soluzione? Non ho sentito - devo dire la verità - parole precise su come sarebbe già oggi possibile provare a ridurre un po' il sovraffollamento attraverso il consolidamento di misure che abbiamo sperimentato e che hanno dato buona prova. Lei sa bene, signor Vice Ministro, che durante gli anni della pandemia abbiamo sperimentato misure alternative nei confronti di coloro che hanno dimostrato di aver svolto con efficacia un percorso di reinserimento: parlo delle misure predisposte per i detenuti a cui sono riconosciute licenze

per i quali sono escluse ragioni di particolare pericolosità. Queste due misure hanno dato buona prova: le abbiamo sperimentate durante la pandemia, le abbiamo prorogate fino al 31 dicembre del 2022 e adesso

siamo in sede di discussione del milleproroghe: dia il Governo parere favorevole agli emendamenti che abbiamo presentato, o almeno si proroghino quelle misure che hanno dato inequivocabile

foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come rilevato dall'interrogante, la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato ad indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia, che alla data di entrata in vigore della legge dispongono ancora di un codice di attività, anche se non detengono animali. La medesima norma ha altresì disposto che, con decreto dell'allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e della transizione ecologica e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo. Lo scorso 30 dicembre, acquisito il concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato emanato il previsto decreto interministeriale: sono ivi stabilite le modalità con le quali i titolari di allevamenti di visoni, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie, da cui ricavarne pelliccia, possono accedere ai benefici economici previsti dalla legge. Il decreto, inoltre, prevede la cessione degli animali, previa sterilizzazione, presso strutture autorizzate ad associazioni animaliste riconosciute e ritenute idonee sulla base di precisi requisiti strutturali e gestionali. Detti requisiti, come pure le modalità di attuazione degli interventi di sterilizzazione,

Rassicuro i senatori interroganti che il decreto contenente le predette disposizioni sarà adottato nei tempi previsti. *(Applausi)*. Signor Presidente ringrazio il Sottosegretario per la risposta e mi ritengo parzialmente soddisfatta, perché era sicuramente importante avere un atto che rendesse effettivamente operativa la normativa, entrata in vigore già da più di un anno. Naturalmente non posso non rimanere attenta e vigile sulla situazione, perché permane, allo stato attuale, un grave rischio per la salute pubblica: lo ha dimostrato quanto verificatosi a Galatea con con l'individuazione di un caso di Covid che ha portato, tra l'altro, all'abbattimento nella struttura degli animali che erano stati contagiati.

quindi, sottolineare quanto i tempi debbano essere i più celeri possibili, proprio per intervenire affinché non si verifichino più casi del genere, nel rispetto anche degli animali, che continuano ad essere stabulati in situazione Per cui, al di là della sofferenza e dello scarso benessere di cui godono in queste piccole gabbie metalliche, è necessario tenere presente anche quanto sia pressante

è la principale arteria stradale di collegamento fra Siena e Firenze, con una estensione di circa 56 chilometri. La sede stradale è costituita da due carreggiate separate, con una larghezza media di 7 metri ciascuna e con due corsie per ogni senso di marcia. Il limite massimo di velocità ordinario è di 90 chilometri ad ora, escluso il tratto dal chilometro 30,500 al chilometro 29,200 direzione Siena, in corrispondenza del viadotto San Giovanni, dove vige il limite massimo di 70 chilometri ad ora. Con riferimento alle rampe di svincolo del tratto in cui sono avvenuti i sinistri stradali causati dai veicoli in transito contromano, la società ANAS ha rappresentato che la segnaletica verticale di accesso è correttamente posizionata. La società ANAS, inoltre, prevede di avviare, nel secondo semestre del corrente anno, una serie di interventi per il potenziamento della segnaletica verticale lungo l'intero raccordo autostradale. Quanto allo stato di riqualificazione del raccordo autostradale 3, sono già attivi ed in fase di attivazione interventi programmati di manutenzione per un importo complessivo di circa 39 milioni di euro. Il MIT è consapevole della gravità del fenomeno dell'accesso in contromano da parte dei conducenti dei veicoli nelle strade a doppia carreggiata, che sovente coinvolgono i veicoli che procedono in senso di marcia regolare. Pertanto, è allo studio un apposito decreto ministeriale per introdurre l'obbligo della segnaletica stradale contromano sulle strade a doppia carreggiata. Con tale provvedimento si intendono definire le caratteristiche della segnaletica verticale ed orizzontale da adottare negli svincoli, nelle intersezioni a raso, nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché negli accessi presenti nelle autostrade e nelle strade a doppia carreggiata. Al fine di rafforzare e di potenziare la segnaletica prevista dal codice della strada e dal regolamento di attuazione si prevede, altresì, l'inserimento del segnale di senso vietato in un pannello fluororifrangente di colore giallo con la scritta ALT, pannello che peraltro è già installato a titolo sperimentale in alcuni punti della rete autostradale, e che verrà installato sia a destra sia a a sinistra di tutte le sezioni stradali esposte al rischio di essere percorse in contromano sulla rete extra urbana stradale e autostradale. Per l'ambito urbano, il potenziamento del segnale di senso vietato sarà realizzato attraverso un raddoppio del segnale stesso sia a destra sia a sinistra della sezione da proteggere. Siffatto provvedimento potrà quindi costituire uno strumento efficace contro il fenomeno del contromano, consentendo anche di aumentare la deterrenza rispetto a condotte di guida pericolose. Signor Presidente, ringrazio il Governo, nella persona del sottosegretario Ferrante. Le risposte che ci ha dato sono altamente positive per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale e delle precauzioni da adottare per evitare questo particolare e tedioso fenomeno, che, come visto, macina vittime in maniera veramente continuativa. Perlopiù, lo spunto di questa interrogazione nasce dal tragico caso di Stefano Sanna, che mi ha dato modo, anche in occasione dell'informativa resa dal ministro Nordio sullo stato della giustizia, di ricordare che il fenomeno della guida in stato di alterazione per l'uso di sostanze alcoliche, così come anche di quelle stupefacenti, costituisce un'altra gravissima situazione che a volte si aggiunge a quella dell'insicurezza delle infrastrutture e che, purtroppo, ha cagionato

ha ricordato di voler intervenire in qualità di Ministro sull'intero *corpus* normativo, per garantire che sulle nostre strade vi siano sicurezza

alle quali risponderanno il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

ha girato sostanzialmente la testa dall'altra parte. Nonostante la ferma opposizione di alcuni Stati, tra cui l'Italia, ha infatti autorizzato l'Irlanda a introdurre, sull'etichetta dei prodotti a base di alcol, indicazioni di carattere sanitario, analogamente a quanto previsto per i prodotti a base di tabacco. La normativa irlandese, infatti, attraverso un messaggio ingiustificatamente allarmistico, equipara il vino e le bevande alcoliche al tabacco. L'adozione di modalità di indicazione sanzionatorie e trasversali come quelle irlandesi fortemente criticata anche dal Parlamento europeo con una precisa risoluzione, a dimostrazione di come la volontà popolare sotto questo aspetto sia chiara e diversa probabilmente da quella di qualche tecnocrate europeo. riteniamo che tale misura sia inaccettabile; lo crediamo noi come Gruppo, ma lo crede anche la maggior parte dell'opinione pubblica italiana nonché i grandi operatori che del vino che hanno fatto di questa Nazione una delle grandi eccellenze, con un valore e un giro d'affari che supera gli 8 miliardi e che ha prodotti riconosciuti per la grandissima qualità. Non si spiega, quindi, perché, se da una parte, i nostri prodotti sono riconosciuti come di grande qualità, dall'altra, vengano penalizzati per una questione - quella sanitaria - utilizzata *ad hoc* solo ed esclusivamente per discriminare alcuni prodotti a vantaggio di altri.

ma la difesa di una maniera di vedere il mondo, e cioè, i prodotti tradizionali contro quello che ormai è evidente a tutti, ovvero il tentativo di discriminare questi prodotti e sostituirli con altri. Le chiediamo, Ministro, come intenda agire per tutelare il diritto del consumatore ad avere anche una corretta informazione, per scongiurare ogni possibile danno a un settore - quello vitivinicolo nazionale - che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale.

questo atto, un tema che riteniamo fondamentale: la tutela della qualità dei nostri prodotti, che viene messa in discussione. È stato ben descritto il quadro nel quale ci muoviamo. La nostra posizione come Governo è netta: qualsiasi etichettatura che preveda uno stigma sugli effetti del vino per la salute umana è inaccettabile. Abbiamo l'impressione che chi lo propone nasconda - dietro l'alto richiamo alla tutela della salute umana - un più pratico intento a impedire ai prodotti di eccellenza italiani, di affermarsi sul proprio mercato. Parliamo infatti di un complesso di obblighi per la creazione di un'etichettatura specifica per i prodotti destinati al mercato irlandese, che potrebbe portare le nostre aziende ad abbandonare quel mercato o a dissuadere gli operatori nel farvi ingresso. Rammento che tutte le misure che impediscono, direttamente o indirettamente, gli scambi presenti o potenziali all'interno dell'Unione europea sono restrizioni vietate dai trattati dell'Unione europea. È per questo motivo che, insieme al vice presidente del Consiglio Tajani, che ha subito sposato la nostra posizione, il 12 gennaio abbiamo inviato una lettera al commissario europeo per il mercato interno Breton denunciando gli effetti distorsivi per il mercato di simili previsioni normative. Non è solo, però, la tutela del mercato che ci interessa, perché è nostra intenzione ristabilire la verità. La misura irlandese non è giustificata da alcuna evidenza scientifica ed è vero, invece, che i rischi per la salute dei consumatori (termine pessimo), delle persone, dipendono dalle modalità di consumo, dal regime alimentare e dallo stile di vita. È una verità che si sposa con gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e che noi riversiamo ai nostri figli, ovvero, che l'abuso di un alimento reca pregiudizio alla salute, non certo il consumo moderato. Vale naturalmente per il vino, ma anche per qualsiasi altro alimento tra quelli ampiamente presenti anche nella dieta dei Paesi nordici. Per queste ragioni è mia intenzione promuovere una serie di iniziative di studio - insieme al Ministro della salute, che mi ha dato ampia disponibilità - sugli effetti del consumo degli alimenti, coinvolgendo i migliori studiosi del nostro Paese, alcuni dei quali, peraltro, hanno già espresso ampiamente le proprie considerazioni, supportate scientificamente in tal senso. Informo inoltre che abbiamo parlato e aperto un canale diplomatico con omologhi di Francia e Spagna, danneggiati anche loro da questo tipo di indicazione, per proporre azioni condivise allo scopo di ribadire la necessità di lavorare sulla distinzione tra consumo responsabile

Non accetteremo mai sistemi di etichettatura degli alimenti che, come il nutri-score, producono effetti discriminatori verso le eccellenze alimentari e noi siamo tra i produttori di eccellenze alimentari -, alterando il mercato e condizionando le persone che vengono definite consumatori finali, ma che noi consideriamo invece detentori della possibilità di scegliere tra prodotti di qualità. Tutto ciò in nome di una informazione corretta e approfondita che intendiamo dare, senza danneggiare le economie e le imprese che a queste sono collegate e che, invece, vanno tutelate proprio difendendo la capacità di discernimento che deve essere garantita alle persone, ai cittadini di tutta Europa e del mondo, ai quali offriamo, attraverso i nostri prodotti non solo eccellenze, ma anche potenziali fattori di benessere.

Sono le *fake news,* come ha detto lei, a nuocere gravemente alla salute, quindi la invitiamo proprio a spingere la ricerca, di concerto con il Ministero della salute, affinché passi il messaggio che è sì importante contrastare l'abuso dell'alcol (lo dico anche da sindaco, perché tante volte veniamo a contatto con chi purtroppo ne abusa), ma che l'uso moderato non solo non è

finestra"). - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: nell'area di sviluppo industriale di Foggia è presente dagli anni '80 del secolo scorso un'importante realtà produttiva, acquisita nel 2019 da G&W Electric Co., primario gruppo statunitense attivo da oltre un secolo nel disegno e nella produzione di prodotti e soluzioni innovative per il settore energetico, che sino ad allora non vantava insediamenti produttivi nel mercato europeo; il ramo di azienda ceduto svolgeva attività di progettazione e produzione di impianti elettrici industriali, contava 120 dipendenti e 20 milioni di fatturato, per il 90 per cento realizzato oltreconfine in più di 40 Paesi; con una comunicazione del 18 febbraio 2022 Confindustria Foggia comunicava alle organizzazioni sindacali e alle competenti autorità pubbliche una nota aziendale con la quale si manifestava la volontà, deliberata il giorno precedente dall'assemblea dei soci della consociata italiana, G&W S.r.l., di mettere in liquidazione la società per perdite; le ragioni addotte sono in parte comprensibili (la recessione collegata alla pandemia, l'aumento dei prezzi e i ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime a livello internazionale), sebbene genericamente addotte, e in parte poco convincenti, laddove si riferiscono ad un'inaspettata quanto necessaria rielaborazione dei prodotti aziendali; la determinazione aziendale comporta la completa cessazione dell'attività, dunque il licenziamento di tutti i 7 dipendenti di Peschiera Borromeo (Milano), nonché di tutti i 114 dipendenti addetti allo stabilimento di Foggia, dei quali ben 69 operai a tempo indeterminato, oltre che dei 13 dipendenti di un'agenzia di somministrazione da sei anni al servizio dell'azienda; molti dei destinatari del licenziamento sono ultracinquantenni e sarebbero di difficile ricollocazione; a far dubitare della fondatezza delle ragioni addotte vi è da un lato l'ampia presenza di personale precario e dall'altro il fatto che nella stessa comunicazione aziendale si indica che i licenziamenti "verranno effettuati nei tempi necessari alla Società per evadere gli ordini già accettati", mostrando come il mercato dei prodotti di questa impresa non sia affatto estinto, come i vertici aziendali avevano sempre riferito alle rappresentanze sindacali;

Foggia lunedì 23 gennaio ha registrato l'indisponibilità totale della parte aziendale nel rivedere la scelta di chiusura; si ritiene sia nella responsabilità del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali intervenire convocando nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico che esplori tutte le possibili

del polo industriale pugliese e milanese. Come si diceva, il complesso aziendale, sorto negli anni Settanta, è stato ceduto nel 2019 a un gruppo statunitense, che fino a ora non risultava avesse esternato alcuna apprensione su una possibile crisi produttiva degli stabilimenti coinvolti, avendo sempre ribadito una buona prospettiva industriale, considerata anche la crescita di lungo periodo dell'intero mercato del comparto elettrico. In data 18 gennaio, invece, per il tramite della Confindustria Foggia, è pervenuta, da parte della G&W all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, una comunicazione ai sensi della legge n. 223 del 1991, riferita al licenziamento collettivo di 114 lavoratori, sette dei quali in servizio presso la sede lombarda di Peschiera Borromeo e gli altri operativi a Foggia, con conseguente cessazione dell'attività. La competente Direzione generale del Ministero mi ha comunicato che allo stato la procedura avviata ai sensi della legge n. 223 del 1991 è in fase sindacale. Sulla questione la Regione Lombardia ha comunicato di non aver avuto ancora comunicazioni ufficiali, ma che metterà a disposizione le azioni di intervento di *moral suasion* a sua disposizione. La Regione Puglia ha invece comunicato che, nelle more dell'eventuale instaurazione presso il il competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* di un tavolo governativo di crisi, il suo comitato di monitoraggio del sistema economico e produttivo delle aree di crisi ha convocato un urgente tavolo regionale di crisi per il prossimo 3 febbraio 2023. Si rassicurano fin d'ora i senatori interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui non dovesse intervenire un auspicato accordo tra i soggetti coinvolti, sarà parte attiva per la costituzione di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e garantisce fin d'ora la disponibilità a lavorare congiuntamente con tutte le parti istituzionali e sociali coinvolte per la salvaguardia, nella misura più ampia possibile, delle attività e dei livelli occupazionali della società oggetto dell'interrogazione.

Signor Ministro, non mi ritengo, per ora, del tutto soddisfatta. Mi permetto di suggerire comunque, vista la presenza di unità produttive pluriregionali e dato il carattere molto specialistico della produzione e la sua destinazione quasi esclusiva verso i mercati esteri, nonché il necessario coinvolgimento di Invitalia per trovare nuovi acquirenti, di attivare un lavoro congiunto della ministra Calderone e dei ministri Urso e Giorgetti.

*(Az-IV-RE)*. Signor Ministro, con questa interrogazione vorremmo avere chiarimenti in merito alla formazione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il tema delle politiche attive ci sta particolarmente a cuore, perché è fondamentale per tantissimi nostri concittadini, ma è anche decisivo per la tenuta del tessuto del nostro sistema produttivo, delle nostre industrie, della manifattura, del vasto mondo dei servizi. È sempre più alta, infatti, la richiesta di manodopera specializzata e il *mismatch*

Questo tema si interseca con l'annuncio che voi avete fatto di una riforma del reddito di cittadinanza ed è su questo punto specifico che vorremmo ascoltare gli intendimenti del Governo. da quello che ognuno di noi pensa sul reddito di cittadinanza, la legge di bilancio stabilisce che i percettori del reddito debbano frequentare per sei mesi un corso di formazione o di riqualificazione professionale. Sarebbe interessante conoscere in quali tempi e con quali modalità il Governo intenda indirizzare questa attività formativa supplementare, anche perché non risulta né che siano state stanziate risorse supplementari, né che ci sia traccia di questi corsi. Tra l'altro, abbiamo letto alcune affermazioni su una presunta intenzione del suo Dicastero di azzerare l'ANPAL, cioè l'Agenzia nazionale che dovrebbe occuparsi di coordinare questa attività. Se così fosse, non ci strapperemmo le vesti, tuttavia forse sarebbe il caso di fare chiarezza anche su questo punto, anche perché abbiamo il timore che l'inazione o la lentezza possano portare ulteriori rinvii rispetto alla riforma del reddito di cittadinanza.

su alcuni obiettivi prioritari dell'azione di Governo in materia di lavoro. Innanzitutto, confermo che è in corso una ricognizione e ritaratura delle funzioni svolte dai soggetti inseriti nella filiera delle politiche attive del lavoro che rivestono ruoli fondamentali come l'ANPAL, rispetto alle quali, però, al momento non è in programma un mutamento di *governance.* Al contrario, il Ministero sta procedendo alle attività normative finalizzate all'aggiornamento dell'assetto statutario dell'Agenzia

Passando al quesito specifico riguardante i percorsi formativi per i percettori del reddito di cittadinanza, voglio sottolineare che con la legge di bilancio il Governo è intervenuto su questo strumento secondo una logica ben precisa, che rappresenta una linea guida per l'azione dell'Esecutivo: rendere la popolazione attiva effettivamente occupabile e sostenerne l'inserimento al lavoro limitando, allo stesso tempo, la possibilità che intere fasce di popolazione siano sostenute esclusivamente attraverso misure di mera assistenza. Considero un obiettivo primario quello di garantire l'attuazione delle norme contenute nella finanziaria e la coerente evoluzione in senso riformatore di quell'intervento. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di frequenza ai corsi di formazione, faccio presente che il programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) già prevede tra i beneficiari i percettori del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l'impiego. Sulla base delle necessità rilevate in sede di valutazione dei bisogni del beneficiario in occasione dell'accesso ai servizi, anche il fruitore del reddito di cittadinanza è pertanto indirizzato in uno dei quattro percorsi previsti per il miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori, tre dei quali prevedono specificamente attività di formazione. Alla data del 31 dicembre 2022, dei 709.127 lavoratori e lavoratrici disoccupati raggiunti e coinvolti dai centri per l'impiego nelle attività del programma, i beneficiari di reddito sono circa 173.000. Si sta intanto procedendo a completare l'attività di presa in carico nell'ambito del programma GOL dei percettori di reddito, con particolare riferimento ai soggetti che ne fruiranno nel corso dell'anno per il periodo di sette mesi. Nel 2023 devono essere assegnate le risorse economiche per una quota aggiuntiva di destinatari programmati, in modo da arrivare, nel 2025, all'obiettivo di 3 milioni di persone raggiunte dal programma GOL, di cui 800.000 coinvolti in attività formative e 300.000 nel rafforzamento delle competenze digitali. In relazione al monitoraggio dei percorsi formativi erogati ai beneficiari del programma GOL, le previsioni della legge di bilancio dispongono lo specifico invio degli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza nel sistema informativo unitario. È prevista a tal fine la registrazione di proposte di aggiornamento e riqualificazione professionale condivise con i lavoratori e il monitoraggio del loro svolgimento. È previsto nell'ambito del comitato direttivo GOL, sede di confronto e decisione tecnica tra Ministero, ANPAL e Regioni, che si predispongano indicazioni operative alla circolare ANPAL n.

attualmente in fase di adeguamento al mutato contesto normativo, si terrà conto di revisionare e creare nuovi strumenti sulla base dei singoli percorsi formativi. Si darà comunque priorità, in coerenza con gli indirizzi europei, alla formazione sulle competenze digitali, soprattutto per giovani e donne, puntando anche alla qualificazione dei percorsi formativi erogati *online* e provvedendo, nel contempo, al monitoraggio della qualità dell'offerta formativa. Concludo, assicurando la massima attenzione sulla tematica segnalata. Il Ministero del lavoro, insieme all'ANPAL, monitorerà l'applicazione delle norme previste nella legge di bilancio, che rappresentano il primo tassello per la costruzione di un nuovo percorso riformatore di inserimento nel mercato del lavoro. A tal proposito, si condivide la posizione espressa dalle senatrici interroganti sulla necessità di introdurre un nuovo modello di inclusione attiva che possa valorizzare e implementare strumenti già sperimentati, rafforzando il percorso di reinserimento e accompagnamento al lavoro.

francamente ci saremmo aspettati una riforma del reddito di cittadinanza già all'interno della legge di bilancio. Così non è stato: avete preferito prendere tempo (circa sette mesi) per realizzare forse più in là la riforma. È vero che ci sono alcuni percettori del reddito di cittadinanza inseriti nel programma GOL, ma leggendo la nota di monitoraggio allo stesso programma risultano non essere superiori al 24,4 per cento (circa 150.000 percettori di reddito). Mi pare che sia una percentuale piuttosto modesta. Con riferimento all'adempimento degli obblighi di istruzione, anche in questo caso mi pare che ci sia un ritardo, perché non risulta che sia stato ancora stipulato il protocollo fra il suo Ministero e il Ministero dell'istruzione. La nostra preoccupazione il nostro timore è che tutto cambi perché nulla cambi, e che accumulando questi ritardi alla fine, anziché trovarci una riforma del reddito di cittadinanza tra qualche mese, voi dobbiate ricorrere all'ennesimo rinvio. E questo sarebbe davvero un peccato per il Paese e per tutti coloro che

La maggiore flessibilità non ha portato maggiore occupazione in unità di lavoro *standard*. Il tasso di occupazione è sempre stato sotto il 60 per cento. Tutti gli obiettivi delle riforme del lavoro, adottate in circa trent'anni, sono falliti. Al contrario, la flessibilità ha portato certamente più precarietà. L'instabilità lavorativa vuol dire anche un incremento notevole di *part-time*, pari addirittura al 46 per cento tra le donne, il dato più alto dell'Unione europea, cento tra gli uomini. Il lavoro a termine è cresciuto negli ultimi due anni, nel periodo di sospensione del decreto dignità, ed ha oggi raggiunto un picco storico di oltre 4,2 milioni di lavoratori: il 22 per cento degli occupati. cento delle posizioni lavorative attive a tempo determinato ha una durata prevista fino a trenta giorni e addirittura il 9,2 per cento di un a risentire di più di questa situazione sono i giovani nella fascia tra i venti e i ventinove anni. Terminata l'emergenza da Covid, il mercato del lavoro appare ancora intrappolato nella precarietà. Il nostro poi è l'unico Paese dell'area OCSE nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale è diminuito invece di aumentare: è infatti diminuito del 2,9 mentre in Germania è cresciuto del 33,7 e in Francia del 31,1 per cento. Nell'insieme, il lavoro atipico rappresenta nel nostro Paese l'83 per cento delle nuove assunzioni. Ripeto: l'83 Il Governo Conte 1, andando in direzione totalmente opposta al *trend* trentennale, aveva adottato il decreto dignità, invertendo la spinta alla flessibilità con un aumento tra il 2018 e 2019 di quasi un milione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Contrariamente a quello che sta avvenendo nel nostro Paese, di recente in Spagna hanno varato una riforma del mercato che permette alle aziende di assumere a scadenza solo in pochi casi previsti per legge, aumentando i lavori a tempo indeterminato del 238 per cento e il tasso di disoccupazione fra gli *under* 25, che aveva toccato il

sociali*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Pirro per i quesiti posti in materia di contratto a tempo determinato e *voucher*. Nell'interrogazione si afferma che le misure di flessibilità, frutto peraltro di scelte politiche ultratrentennali e di varia colorazione politica, abbiano significato aumento della precarietà, contratti di lavoro di durata particolarmente limitata e con retribuzioni inadeguate, oltre che un diffuso uso del *part-time*. Al contrario, il cosiddetto decreto dignità avrebbe rappresentato un argine al modello di precarietà. In realtà, le norme che cita come strumenti di tutela del lavoratore hanno incentivato una generalizzata riduzione della durata dei contratti a tempo determinato, dal momento che il decreto dignità ha previsto che i contratti a termine potessero essere privi di causali se di durata fino a dodici mesi. Rammento poi che è stato anche il Governo Conte, con il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto rilancio, per esigenze legate alla crisi pandemica, a prevedere la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i cosiddetti contratti a tempo determinato acausali, ossia i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato privi di condizioni. Sulla stessa materia è poi intervenuto il cosiddetto decreto sostegni, il decreto-legge n. 41 del 2021. Flessibilità e precarietà non sono concetti equivalenti, soprattutto perché credo che la prima rappresenti la capacità di adattarsi efficacemente e adeguatamente alle esigenze economico-sociali contingenti, fossero anche quelle emergenziali o straordinarie, che ci auguriamo non dover più vivere. La flessibilità, insomma, è necessaria, perché consente a imprese e lavoratori di uniformarsi alle molteplici e variabili situazioni di mercato e alle sfide globali cui le comunità sono chiamate a fare fronte e impongono forme flessibili di lavoro che siano adeguate e funzionali agli obiettivi da raggiungere. Non è mia intenzione eliminare ogni tipo di causale dai contratti a tempo determinato e lo riaffermo in questa sede. Allo stesso modo, credo che una rigida tipizzazione legale delle causali dei contratti a tempo determinato possa rappresentare un limite per il sistema imprenditoriale e lavorativo del Paese. Mi impegno quindi a rivedere l'istituto del contratto a termine per precisarne i contenuti, renderlo uno strumento efficace ed elastico di incremento dell'occupazione e prevederne limiti tali da garantire un maggior controllo della legittimità del suo utilizzo. Ritengo anche che sia preferibile l'opzione di demandare alla contrattazione collettiva l'indicazione delle causali che legittimano l'utilizzo di questo istituto. Nell'interrogazione si fa un generico riferimento anche allo strumento dei *voucher.* Ricordo che lo strumento risale alla cosiddetta legge Biagi del 2003, nel cui impianto normativo originario, più volte integrato

uno spazio occupazionale nuovo. Premesso, quindi, che i *voucher* non sono certamente uno strumento introdotto da questo Governo, come pure lascia pensare l'interrogazione, non condivido in ogni caso la conclusione che questi siano uno strumento che necessariamente stimola il precariato. In talune occasioni, in relazione alle esigenze delle famiglie, essi possono permettere di dare una base giuridica per retribuire attività saltuarie, quali piccoli lavori domestici o l'insegnamento privato supplementare. Un ulteriore esempio delle finalità positive degli interventi assunti in materia con la legge di bilancio è rappresentato dal *voucher* agricolo, che con l'ultima legge di bilancio è stato disciplinato in maniera rigorosa e precisa, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. Il *voucher* agricolo è un istituto diverso dal *voucher* previsto dalla legge Biagi, in quanto si tratta di una prestazione di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, dove vengono assicurate ai lavoratori ampie tutele. Il suo utilizzo è consentito ai soli datori di lavoro che rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso è determinato sulla base dei livelli retributivi stabiliti dal contratto collettivo di settore ed è fissato un limite massimo di durata delle prestazioni di quarantacinque giorni all'anno. *(M5S)*. Signor Ministro, purtroppo non sono affatto soddisfatta delle risposte. Mi domando come si possa dire che il decreto dignità non sia stato efficace e abbia aumentato la precarietà quando, in realtà, ha portato a un milione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, riducendo parimenti quelli a tempo determinato. Esso introduceva delle causali che giustificavano l'attivazione dei contratti a termine, non abolendoli, ma appunto solo con determinate motivazioni, esattamente come sta avvenendo in Spagna, con i risultati ottimi che le ho già citato. Sulla questione dei *voucher*, che non esistevano più - quindi li avete, di fatto, reintrodotti o introdotti - non mi soffermo sul fatto che le famiglie avevano già degli strumenti a disposizione adeguati, come il libretto famiglia, per regolarizzare i propri collaboratori. Inoltre, il *voucher*, così come è stato introdotto in agricoltura, può prestarsi facilmente ad abusi e al lavoro nero. L'ultimo punto che mi permetto di sottolineare è che martedì è venuta in audizione in 10ª Commissione

contratti di un giorno e poi rimangono settimane a casa, poi lavorano di nuovo due giorni o una settimana, quando mai potranno pensare seriamente di staccarsi dal nucleo familiare di origine, creare una propria famiglia e mettere al mondo dei figli in una situazione così precaria? Allora, se volete essere il Governo della famiglia e dell'aumento della natalità del nostro Paese, forse il punto*...

chiaramente di misure nate in epoca Covid, ma sappiamo che quest'epoca non ce la siamo lasciata completamente alle spalle e che le ultime rilevazioni mostrano un incremento dei contagi che impone la necessità di mantenere alto il livello delle misure preventive. preventive. Succede ora che nella vostra legge di bilancio, al comma 306, prorogate alcune di queste misure. Si dice che il datore di lavoro dovrà assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile alle categorie di lavoratori in questione, ma sembra - è stato evidenziato anche dal Servizio studi del Senato - che la formulazione di questa nuova norma transitoria - come dicevo, è al comma 306 - non contempli il caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità

una serie di lavoratori rimane nel limbo dell'incertezza, svolgendo delle funzioni che non sono compatibili con quelle del lavoro agile: pensiamo agli infermieri, ai medici, a una serie di operatori sanitari, quelli cui tutto il Parlamento applaude per il grande lavoro e il sacrificio che hanno fatto, salvo poi dimenticarsi che esistono e metterli quindi in sicurezza. Abbiamo provato ad aiutare il Governo e glielo dico perché nel decreto proroga termini in

Condivido la considerazione che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile raggiunga uno scopo importante a tutela dei lavoratori più vulnerabili attraverso la funzione di protezione e, soprattutto, di inclusione socio-lavorativa delle diversità. Per questo motivo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sosterrà ogni iniziativa volta alla proroga almeno trimestrale dello strumento, al fine di proseguire nell'azione di protezione dei soggetti più esposti al rischio della malattia da Covid-19. Sul punto assicuro che è già in corso un'interlocuzione tecnica con i competenti uffici del Ministero per la pubblica amministrazione per la valutazione congiunta degli interventi normativi necessari, ma daremo parere favorevole.

di conversione, sentirò il Governo dare parere favorevole agli emendamenti del Partito Democratico e a quel punto immagino che ci sarà il voto unanime di tutta la Commissione.

e che poi si sono dimenticate alla prova dei fatti di realizzare, come stiamo vedendo anche in questi giorni. Spesso ci sentiamo rispondere che è un programma di legislatura, per cui sono necessari almeno cinque anni. Quello che noi vi diciamo è che c'è una serie di emergenze e i lavoratori fragili sono un'emergenza. Ve li siete dimenticati. Siamo contenti se abbiamo potuto aiutarvi a costruire in modo migliore una norma che potrà andare in aiuto a tante famiglie e a tanti lavoratori che si trovano in difficoltà.

Signor Presidente, colleghi, pongo oggi all'attenzione dell'Assemblea e del Governo, autorevolmente rappresentato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ringrazio, la questione delle infrastrutture e in modo particolare della strada provinciale 47 della Valsugana, che collega Padova a Cittadella, ricordando che il tratto da Cittadella a Bassano e da Bassano a Trento è già strada statale. di un'opera essenziale di collegamento tra l'Italia e tutto il Nord Europa: ci tengo a sottolinearlo, perché sono consapevole dell'importanza che il ministro Salvini ha da sempre rivolto alla necessità, per il nostro Paese, di essere competitivo rispetto anche agli altri Stati. Nella provincia di Padova, cuore produttivo del Nordest, ci sono circa 76.000 imprese. Da oltre dieci anni i sindaci dei Comuni dell'alta-padovana, i cittadini e il mondo produttivo attendono che venga realizzato un moderno collegamento viario in una delle aree più urbanizzate e industrializzate del Veneto e d'Italia. Ritengo essenziale intervenire per potenziare l'intero sistema viario della provincia di Padova e chiaramente del Veneto. In questa sede mi limito a evidenziare l'importanza dei corridoi viari tra la provincia di Padova e la superstrada Pedemontana veneta. Ci sono due corridoi naturali: quello della strada regionale 308, Strada del Santo, e la strada provinciale 47 della Valsugana, che può essere una chiave di accesso del Nord-Est alla Pedemontana veneta e - come dicevo prima - alle principali infrastrutture di comunicazione. Lo sviluppo socio-economico - come tutti sappiamo - non può prescindere dalle infrastrutture viarie e tecnologiche che si realizzeranno nei prossimi anni. Parliamo di un territorio che non può rimanere escluso dai principali corridoi corridoi commerciali europei. Ecco perché, cogliendo le richieste degli amministratori locali, del territorio e dei rappresentanti delle categorie economiche, ho deciso di sottoporre oggi la questione all'attenzione del Ministro. Chiedo pertanto al Governo il passaggio del tratto della strada provinciale 47, tra Padova e Cittadella, a strada statale, e quindi sotto la gestione dell'ANAS, così da permettere il mantenimento e soprattutto, *in primis*, l'adeguamento della strada in arteria a scorrimento veloce e il suo collegamento con la superstrada Pedemontana

onorevoli colleghi, approfitto, visto che partiamo dal Veneto, per ricordare l'amico Paolo Saviane e salutare Daniela e Beatrice, con cui abbiamo condiviso tanti impegni in quest'Aula e a cui dedichiamo buona

quando siamo al Governo, e penso che la direzione da lei indicata sia quella giusta, e non solo per questa strada, ma anche per altre. Concordo con lei sulla rilevanza delle piccole arterie, perché contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del tessuto economico e sociale e a migliorare la mobilità dei cittadini. Proprio in considerazione di tali aspetti, il tratto della provinciale 47 della Valsugana, che collega Padova a Cittadella, è rientrato nella proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale presentata dalla Regione Veneto, che in passato ha avuto qualche lungaggine di troppo, ma penso che in questi novantasette giorni abbia avuto una sostanziale e sostanziosa accelerata. Su tale proposta, infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere positivo nel novembre scorso. Stiamo ora predisponendo gli atti per l'acquisizione della prescritta intesa nella prima seduta utile della Conferenza unificata. Successivamente, con l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di viabilità - lei sicuramente avrà modo di accompagnare - concluderemo positivamente l'*iter* procedurale con l'emanazione del relativo DPCM. Aggiungeremo così un ulteriore tassello allo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese per poter giungere al completamento e al potenziamento della strada in argomento, attraverso il suo adeguamento in arteria a scorrimento veloce e il suo collegamento con la superstrada Pedemontana veneta. In sostanza, se la Provincia e la Regione ritengono che lo Stato possa gestire meglio questa arteria, lo facciamo e ne siamo contenti. Altro paio di maniche è la riforma - dal mio punto di vista si rivelerà necessaria - di reintrodurre le Province elette direttamente dai cittadini, con personale, competenze, denari e poteri per tornare a fare quello che le Province hanno brillantemente fatto per tanto tempo.

Fino ad oggi, però, non è stato possibile completarla, perché la Provincia autonoma di Trento, nonostante siano passati cinquant'anni, per tanto tempo non ha individuato quello che era l'innesto a Nord, appunto, della Valdastico. Ora, c'è una novità - ed è il motivo per cui oggi la interrogo - nel senso che Trento ha individuato la soluzione a suo giudizio più idonea, che è quella di un innesto in prossimità di Rovereto Sud. È sufficiente consultare una cartina geografica, Ministro - lei lo avrà fatto sicuramente - per capire che questa, forse, non è la soluzione più razionale; però, da autonomisti che rispettano, dal punto di vista non solo costituzionale ma anche morale,

il collega De Poli parlava della Valsugana - che verrebbe sicuramente alleggerita di molto: la famosa Pedemontana veneta avrebbe uno sbocco a Nord e i prodotti delle nostre imprese vicentine, venete avrebbero un innesto diretto verso i grandi mercati del Nord Europa.

la decisione di completare a Nord l'autostrada Valdastico; cosa pensa lei, Ministro, dello sbocco a Rovereto Sud ipotizzato dalla Provincia di Trento, e quali iniziative intenda assumere il suo Dicastero per arrivare al completamento a Nord dell'infrastruttura. Da ultimo, le pongo una domanda forse un po' più complicata. Io le chiederei di smentire, signor Ministro, quelle quelle note apparse sulla stampa, secondo cui un certo tergiversare nell'*iter* di completamento a Nord dell'autostrada sia finalizzato ad arrivare alla revoca della concessione. Questa è un'ipotesi che io reputo, anche da avvocato, piuttosto complicata e che potrebbe portare a dei contenziosi che poi allontanerebbero troppo nel tempo l'opportunità che oggi abbiamo di completare a Nord

il Ministro ascolta il presidente Fugatti e il governatore Zaia. È chiaro che stiamo valutando i flussi di traffico e stiamo ascoltando i territori. A proposito del Vicentino c'è il tema della bretella, su cui ci stiamo confrontando col sindaco di Vicenza, perché

del ragionamento che andrò a svolgere, partendo dalla fine. Sulla convenzione relativa all'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova è già stata avviata la procedura di revisione, sulla quale attendiamo un riscontro della Commissione europea. quindi la norma; già ho ereditato il problema dell'Autostrada dei parchi A24-A25, altri contenziosi non ne desidererei. Il senatore ha ricostruito la vicenda di questa avveniristica ne ho parlato poco tempo fa con il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ho sentito anche questa mattina, come ho sentito l'assessore De Berti; abbiamo concordato sulla necessità di avviare un confronto definitivo per arrivare alla scelta conclusiva. In sostanza, l'ascolto e la condivisione dei territori è fondamentale, ma secondo lo stesso codice dei contratti, che quest'Assemblea dovrà approvare entro il 31 marzo, la politica dovrà prendersi l'onore e l'onere di scegliere. Ad esempio, il codice dei contratti prevede il superamento del dissenso

altrimenti mi assumerò l'onore e l'onere di dare alle imprese, ai territori e alle istituzioni venete e trentine una via di soluzione. la via che mette d'accordo tutti. Se non ci sarà, su questa come su altre grandi infrastrutture, può contare sul fatto che alla fine mi prenderò la responsabilità di prendere la decisione in tempi celeri.

tutte le sue caratteristiche la rendano un uomo di decisione, con capacità di prendere decisioni, un decisionista. Da questo punto di vista non posso che ricordare le parole del nostro presidente Berlusconi, secondo cui noi uomini del centrodestra siamo uomini del fare e vogliamo che i problemi vengono risolti.

nazionale, ma anche del territorio. Nelle prossime settimane a Vicenza si terranno le elezioni provinciali; probabilmente anche una pronuncia del nuovo Presidente della Provincia su questo tema la può aiutare nella sua decisione. Mi dichiaro quindi

Alcune di quelle infrastrutture presentano fragilità strutturali e sono ormai chiuse perennemente al traffico pesante: è il caso, in particolare, del ponte tra i Comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, un'infrastruttura viaria d'importanza cruciale per il sistema dei collegamenti e della mobilità nei territori lombardo-emiliani. Purtroppo i lavori per la sua realizzazione sono in corso da anni e non è ancora chiara la data di ultimazione. L'attuale ponte fu realizzato negli anni Sessanta e da allora ha subito numerose ristrutturazioni. Il sisma del 2012 ha indebolito irrimediabilmente la struttura ed è stato inevitabile il nuovo blocco del traffico pesante, regolato tramite strettoie agli accessi. Queste limitazioni sono presenti da anni, creando un disagio insostenibile alle comunità locali. Nel settembre 2013 sono iniziati gli studi del progetto per il nuovo ponte per la parte in alveo; la fine dei lavori era prevista per l'inizio del 2019. Oggi però il ponte è realizzato solo parzialmente. Dopo tanti anni, quindi, ci troviamo davanti al rischio di indizione di una nuova gara, che comporterebbe un aggravio di quattro o cinque anni minimi, necessari per finire i lavori; a ciò si aggiungono gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con un ulteriore incremento del quadro economico complessivo dell'opera. Nella stessa Provincia, anche il ponte tra Ostiglia e Revere, infrastruttura in parte ferroviaria e in parte stradale, attende ormai da diversi anni lo sblocco della progettazione e lo stanziamento delle risorse. Nella scorsa legislatura, grazie a un emendamento del Gruppo Lega, si è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, da utilizzare, da parte delle Province territorialmente competenti e dall'ANAS, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione e il completamento di nuovi ponti nel bacino del Po. Signor Ministro, si chiede di sapere e quali iniziative di sua competenza intende assumere al fine di accelerare le procedure di manutenzione e, ove necessario, di ricostruzione dei ponti sul fiume Po, anche in relazione al fondo che ho appena citato.

perché leggere i documenti su carta è un conto, andare sui ponti e incontrare i sindaci, le comunità e le associazioni gli imprenditori è un altro paio di maniche. Nello scorso fine settimana ho visitato le Province di Mantova, di Cremona e Pavia. La messa in sicurezza delle migliaia di ponti e viadotti, che in alcuni casi cinquant'anni di vita sulle spalle, è una mia priorità. Per quello che riguarda il ponte di cui lei parlava, su cui è vietato il transito - ahimè da troppo tempo - degli autobus e dei mezzi pesanti, con tutto quello che ne consegue, il mio Ministero ha in previsione due modifiche normative per arrivare alla procedura negoziata diretta per l'assegnazione dei lavori. Stiamo reperendo anche i milioni necessari che sono sopraggiunti per l'incremento delle materie prime. Mi sono ripromesso di arrivare, entro l'estate, all'apertura almeno al traffico leggero del ponte di San Benedetto. Il ponte di Ostiglia ha avuto la ventura, proprio nei giorni scorsi, di ricevere l'autorizzazione per la società ANAS di acquisire da RFI la rete ferroviaria, che non verrà più utilizzata e che diventerà una parte del ponte. Su questo si stanno reperendo i fondi necessari, anche grazie ai contributi che i Gruppi Lega in passato sono riusciti a a mettere da parte. Ne approfitto per passare da Mantova a Pavia (sempre bassa lombarda). Ho visitato anche la Provincia di Pavia e confermo che abbiamo trovato i 7 milioni necessari, deliberati dal CIPES nello scorso dicembre, per il ponte di Vigevano, che dovrà essere la conclusione della Vigevano-Malpensa, di cui si parla da alcuni decenni. Così come un altro ponte, il ponte della Becca, ha fatto passi avanti: la Provincia di Pavia ha già redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica e ha indetto la conferenza dei servizi preliminare, alla cui conclusione il progetto sarà trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovverosia arriverà al mio Ministero, per l'acquisizione del prescritto parere. Assicuro che lavoreremo speditamente per portare avanti anche questa opera fondamentale, non solo per la Provincia di Pavia. Su un altro ponte, di cui si parla da alcuni decenni e per le cui parole gli italiani hanno già speso circa 300 milioni di euro, un po' più a Sud, le posso assicurare che stiamo lavorando con determinazione e coraggio e che entro due anni poseremo la prima pietra.

in particolar modo della Provincia di Mantova. Quella del ponte di San Benedetto è una storia lunga che ha creato e sta creando molto disagio e anche danni economici incalcolabili alla Provincia di Mantova. Sono molte le aziende che hanno perso ordinativi, alcune hanno dovuto chiudere, alcune hanno dovuto delocalizzare il sito produttivo. Ma oltre al danno economico c'è anche il danno sociale. Il territorio di Mantova è esclusivamente pianeggiante. Il Comune di San Benedetto dista dal Comune capoluogo 25 chilometri. Il danno sociale è che alcuni ragazzi, per poter

risposta, signor Ministro. Lei è una persona determinata: sblocchi definitivamente la situazione e risolva questi problemi anche tramite il nuovo codice degli appalti, un codice che velocizzi l'*iter* di realizzazione e completamento delle opere e non le blocchi. Le auguro buona fortuna e buon lavoro.